«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19» Comunico che in data 9 giugno 2021 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri per la pubblica amministrazione e della giustizia* «Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazione di ripresa e resilienza

Signor Presidente, visto il poco tempo per illustrare la mozione, cercherò di entrare subito nel merito, partendo dai punti che riteniamo essenziali per chiarire le motivazioni per cui abbiamo presentato l'atto di Nel gennaio 2021 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha dichiarato le larve delle tarme della farina sicure per il consumo umano; il 3 maggio scorso i Paesi membri dell'Unione europea hanno approvato una proposta della Commissione per autorizzare la commercializzazione delle larve come ingrediente di altri alimenti.

isolati o prodotti a partire da colture cellulari o colture di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe costituiscono una delle categorie di nuovi alimenti elencate nel regolamento;

entro fine del 2022 un'etichettatura nutrizionale armonizzata e obbligatoria a livello europeo da posizionare sulla parte e, tra le varie tipologie di etichettatura alimentare sperimentate e sviluppate all'interno dell'Unione europea, si è profilata l'ipotesi di adottare il cosiddetto «Nutri-score»;

immateriale dell'umanità dall'UNESCO, trattandosi di uno stile di vita particolare, che - leggo testualmente - «comprende una serie di competenze, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni concernenti la coltivazione, la raccolta, la pesca, l'allevamento, la conservazione, la cucina e soprattutto la condivisione e il consumo di cibo». In pratica, è la nostra identità nazionale. Non abbiamo presentato questa mozione in maniera estemporanea, ma è un lavoro che proviene da lontano. L'abbiamo voluto ricordare all'interno della stessa mozione, mozione, citando che il 12 febbraio del 2020 è stata approvata alla Camera dei deputati, all'unanimità, una mozione d'iniziativa del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia, che evidenziava i rilevanti dubbi, sia di carattere scientifico sia di ordine economico, inerenti a tale sistema e impegnava il Governo ad adoperarsi in sede europea per contrastare l'adozione del nutri-score e tutelare il settore agroalimentare italiano.

valorizzare e promuovere le eccellenze agroalimentari di produzione italiana; adottare tutte le iniziative necessarie per difendere il prodotto vitivinicolo italiano e i prodotti DOCG, DOC e IGT; adottare le opportune iniziative per evitare di chiamare carne quello che non lo è; è; dare ai nostri produttori agroalimentari più adeguati strumenti per difendersi dall'*italian sounding,* pratica commerciale che riteniamo sleale, al pari della contraffazione, e, contestualmente, maggiori risorse per promuovere i prodotti italiani; contrastare, in maniera ferma, in sede europea, ipotesi di adozione del nutri-score o del sistema a semaforo, ribadendo la contrarietà dell'Italia ad ogni sua forma di applicazione e contemporaneamente sostenere invece il nutrinform battery, che risulta essere un modello di etichettatura maggiormente efficace e più affine alla tutela della dieta mediterranea; prevedere una campagna informativa su questo nuovo sistema di etichettatura proposto dall'Italia, che permetta ai consumatori di avere informazioni nutrizionali chiare e precise e prevedere una fase di sperimentazione temporanea di questo tipo di etichettatura su tutto il territorio nazionale, attraverso incentivi alle imprese che utilizzino il nuovo marchio. Tutto questo, in sintesi, è la mozione a prima firma del collega De Carlo, con cui Fratelli d'Italia chiede a quest'Assemblea un voto unanime e condiviso a difesa dell'agroalimentare italiano. *(Applausi)*.

affinavano sempre di più principi di difesa da marchi contraffatti e la promozione del nostro settore agroalimentare, che rappresenta un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale. Ad esempio, la legge n. 80 del 2005 rafforzò la tutela giuridica del marchio "*Made in Italy*", estendendo le sanzioni contenute nella legge finanziaria 2004, che si limitava alle false e fallaci indicazioni di provenienza anche alle indicazioni di origine; l'uso improprio del marchio e la sua contraffazione sono quindi sanzionati penalmente con ammende e, in alcuni casi, con l'arresto. La legge n. 166 del 2009 poi introdusse il nuovo marchio di origine, il "100 per cento a vantaggio delle imprese che hanno mantenuto la produzione sul territorio italiano senza ricorrere alla delocalizzazione. Alla luce di quanto detto, è evidente che già la normativa tenda a contrastare i fenomeni di plagio o contraffazione del prodotto italiano. Il settore agroalimentare, che rappresenta una quota rilevante delle esportazioni del nostro Paese, è un ambito nel quale il *made in Italy* è sinonimo di alta qualità del prodotto e per tali ragioni la contraffazione assume proporzioni rilevanti. Tale garanzia di fiducia non può ridursi alla semplicistica comunicazione grafica, che certamente potrebbe risultare più semplice e immediata nella lettura, ma limiterebbe l'interpretazione del consumatore sugli apporti nutrizionali dei singoli alimenti. D'altro canto, l'impegno del nostro Paese è sempre stato orientato alla massima trasparenza sull'indicazione di origine in etichetta per tutelare i consumatori più virtuosi e garantire il diritto dei consumatori a una corretta informazione. Questa non può però essere riduttiva e limitativa, pregiudicando la capacità di diffondere informazioni sui nutrienti degli alimenti, andando a sminuire l'intelligibilità da parte del consumatore. Il nutri-score, che è il sistema di etichettatura dei prodotti alimentari sviluppato in Francia dal 2016 e che si avvale, in maniera impropria e fuorviante, dell'utilizzo di una scala cromatica e di una alfabetica per la classificazione dei valori nutrizionali di un prodotto alimentare, si pone apertamente in contrapposizione con i principi della dieta mediterranea, che invero si fonda su un consumo bilanciato di tutti i nutrienti. Una simile impostazione penalizzerebbe fortemente le produzioni agroalimentari nazionali, gli alimenti tradizionali e altamente salutari come, ad esempio, l'olio extravergine d'oliva e numerose produzioni DOP e IGP, che riceverebbero una valutazione negativa tradotta in un bollino rosso per via del loro contenuto di sale, zuccheri e grassi. Al riguardo, l'Italia ha avanzato una proposta alternativa, il cosiddetto schema a batteria, ribadendo che simili modelli devono restare volontari e non obbligatori ed escludendo da un'eventuale applicazione obbligatoria le produzioni a indicazione geografica. Questo schema, anche noto come nutrinform battery, indica al consumatore i valori nutrizionali dell'alimento in rapporto al relativo fabbisogno giornaliero e al corretto stile alimentare. Le dette diciture peraltro avrebbero carattere aggiuntivo e non sostituirebbero la classica etichetta nutrizionale posta sul retro della confezione. Altre tecnologie verrebbero incontro alle esigenze dei consumatori, come la *blockchain*, che permetterebbe la piena tracciabilità alimentare, fornendo dettagli d'origine sulle materie prime, informazioni su produzione e lavorazione, date di stoccaggio e spedizione dei vari prodotti. Tale tecnologia, per le sue peculiari caratteristiche, andrebbe sempre più promossa a tutela delle produzioni e dei marchi tipici per certificare l'origine degli alimenti, che è storia di donne, di uomini e della loro cultura, nonché di territori e delle loro tradizioni e che riconquisterebbe così la fiducia dei consumatori. L'augurio è che una maggiore semplificazione, trasparenza e tutela del marchio d'origine a vantaggio dei consumatori e delle piccole e medie imprese,

politiche a sostegno della qualità e delle caratteristiche intrinseche delle produzioni agroalimentari nazionali, nonché dell'esattezza e della veridicità dei dati riportati in etichetta, intensificando la lotta contro le frodi alimentari e incoraggiando una corretta educazione alimentare. Concludo affermando che la promozione e la diffusione della dieta mediterranea quale modello sostenibile da un punto di vista alimentare, produttivo e ambientale devono essere il traino per la salvaguardia della biodiversità e per il sostegno di politiche a tutela del lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura. Signor Presidente, colleghi senatori e senatrici, signor Ministro, ancora una volta ci troviamo a discutere in Assemblea di *made in Italy*, in questo caso dell'agroalimentare italiano, quella filiera terra-cibo-tavola che rappresenta il 25 per cento del PIL del Paese, che nel 2020, con 46 miliardi di euro, ha segnato un incremento dell'1,9 per cento, a conferma che agricoltura e agroalimentare italiani, oltre ad essere stati pietra miliare dell'economia passata, sono fattori strategici per l'economia presente e futura. Come già ho avuto modo di dire, i prodotti italiani sono eccellenze che tutto il mondo ci invidia, coltivate, lavorate e conservate in contesti territoriali caratterizzati da Nord a Sud da una miriade di situazioni di microclima. Non vi è prodotto, fra le migliaia, che risulti uguale, spostandosi nei nostri meravigliosi territori, con sapori, profumi e gusti invidiati in tutto il mondo. Da qui nascono i sabotaggi, la concorrenza sleale, il gioco sporco e l'*italian sounding* agroalimentare - che chiamo lo scimmiottamento del *made in Italy*, che va dall'imitazione a etichettature o immagini ingannevoli, se non contraffatte il sistema a semaforo nutri-score, che alcuni Paesi vorrebbero far adottare per affibbiare impropriamente il colore rosso alle eccellenze italiane e a prodotti della nostra dieta mediterranea, che pure

Ecco appunto i missili puntati sui nostri prodotti buoni, sani e salutari, che tentano di colpire il nostro Paese: i cibi sintetici, le non carni e il non latte vegetali o le proteine di vermi. vermi. Lega Salvini Premier-Partito sardo d'Azione cosa chiede quindi con questa mozione? Chiede un impegno del Governo nelle seguenti direzioni: ad adoperarsi in tutte le opportune sedi per contrastare qualsiasi iniziativa discriminatoria nei confronti del modello alimentare basato sui principi della dieta mediterranea e per difendere la salute dei consumatori da sistemi di etichettatura fuorvianti e ingannevoli, al fine di tutelare il nostro patrimonio agroalimentare; ad agire in linea con i contenuti del disegno di legge n. 1060, recante disposizioni volte a incentivare il raggiungimento di *standard* qualitativi elevati dei prodotti agroalimentari italiani, introducendo un sistema di *rating* per la certificazione di eccellenza e riforma del sistema di prevenzione, al fine di migliorare la trasparenza sull'etichettatura con l'obiettivo di far conoscere le forti criticità del nutri-score e apportarvi le conseguenti dovute correzioni; puntare su obiettivi strategici nella progettualità del PNRR; a migliorare la salute dei cittadini, tutelando i consumatori in materia di composizione degli alimenti e privilegiando la salubrità e i cambiamenti dei modelli di consumo, orientati a benessere e longevità; a promuovere le nostre eccellenze, correggendo le storture del nutri-score, nonché un indice di scala intuitivo, non a colori, che permetta ai consumatori una maggiore consapevolezza di ciò che mangiano, secondo i principi di qualità e salubrità, che non possono essere a basso costo; ad assumere ogni iniziativa a livello europeo affinché venga accolta una

da un altro gruppo politico, ma sui *media* è passato che solo quel gruppo politico, che non menzionerò, ha a cuore la difesa del *made in Italy* agroalimentare. Così non si fa: su questo tema bisogna essere uniti le bandierine non portano niente di buono. Non porta niente di buono nemmeno fare questa battaglia solo in Italia. Questa battaglia si fa per lo meno in Europa,

restiamo come siamo rimasti finora. Chiunque possa partecipare a una fiera agroalimentare, ad esempio la Anuga (che è la più grande del mondo), può vedere che accanto allo *stand* ICE o di qualche produttore italiano ce ne sono dieci tedeschi o cinesi di *made in Italy* o di *italian sounding.* Dobbiamo capire che il campo da gioco è l'Europa e quindi o siamo europeisti non per scelta fideistica e impariamo a esserlo in modo efficiente, oppure siamo dei provinciali e il risultato si vede.

Dopo dieci anni di battaglie sono riuscito a ottenere, insieme ad altri colleghi, questo riconoscimento, ma da sei mesi manca il decreto di attuazione. La ristorazione italiana all'estero è il primo difensore e promotrice del *made in Italy* agroalimentare. Nella legge che almeno il 50 per cento dei prodotti serviti nelle catene di veri ristoranti italiani all'estero siano DOP, DOC e IGT, ufficialmente riconosciuti dall'Unione europea come prodotti di eccellenza italiani. Perché poi non utilizziamo

altrimenti non sarebbero state presentate ben cinque mozioni sull'argomento. Tuttavia, credo di poter dire che ciascuno di noi ha interesse per il mondo delle produzioni italiane.

Per questo è essenziale che in Europa si trovino alleanze e che non si alzino muri, come invece forse qualcuno intenderebbe fare. Alla chiusura rispetto al dialogo e al confronto non corrisponde mai nessuna promozione: credo che questo lo dobbiamo avere chiaro e la nostra mozione lo mette in risalto.

quanto il prodotto italiano e in particolare la cultura, la storia e la composizione delle nostre diete e dei nostri prodotti siano fondamentali anche per il benessere. Ormai è riconosciuto, non diciamo niente di nuovo

ha anche benessere dal punto di vista della salute. È per questo che anche i Ministeri lavorano insieme. È già stato affrontato da chi ha presentato la mozione il tema dell'etichettatura

già stato detto, invitiamo il Governo a farsi promotore in Europa del fatto che il nutri-score venga abbandonato come sistema e che si diano invece campo, gambe e forza ad altri sistemi che garantiscano al meglio l'informazione del consumatore e quindi

avvio a concludere, ribadendo ancora quanto già detto rispetto al fatto che c'è davvero la necessità di confrontarsi in sede europea

Credo che lo faremo soltanto facendo capire a tutti i Paesi, anche a quelli più vicini, che non vogliamo conquistare il mondo, ma ne avremmo tutto il diritto e che soprattutto, da parte dell'Italia, si può imparare come fare bene per formare, educare e promuovere il prodotto e un'alimentazione sana e di qualità. Signor Presidente, gentili colleghi e colleghe, Ministro, le mozioni in esame ci danno l'opportunità di precisare determinate situazioni, perché sembra che qui il mondo vada all'incontrario. In Europa, in campo alimentare, sta prendendo sempre più piede una politica che sembra proprio minare la qualità agroalimentare dell'Italia. Lo vediamo con l'introduzione, nella nostra cultura alimentare, di alcuni alimenti che non ne fanno parte, tipo la farina degli insetti o il vino dealcolizzato. se vogliamo parlare di alimentazione sana, dobbiamo necessariamente ricorrere al concetto della dieta mediterranea, che non è tanto un insieme e un elenco di alimenti, ma è uno stile di vita. Quell'educazione alimentare che noi abbiamo portato anche nelle scuole, per la formazione dell'individuo e del bambino, deve essere riconosciuta e non deve essere assolutamente messa in discussione, anche attraverso dei meccanismi che a questo punto definirei perversi, come il nutri-score, che va a determinare la salubrità di un elemento solamente con dei colori, non inserendolo in un prospetto di dieta alimentare che necessariamente deve riferirsi al consumo giornaliero e addirittura settimanale di determinati alimenti. Ecco che, così facendo, si introducono alimenti

Veronesi - che va a combattere malattie come il diabete, l'ipertensione e anche malattie neurovegetative (parliamo dell'Alzheimer e del Parkinson). Attraverso il meccanismo perverso del nutri-score troviamo alimenti preziosissimi per la nostra salute - voglio fare l'esempio dell'olio d'oliva - che classificati, su quella scala di colori, come alimenti non eccellenti. Il nutri-score va a coinvolgere anche le eccellenze del nostro agroalimentare, l'IGP e il DOP. Naturalmente è stato fatto un lavoro rispetto a questo meccanismo,

andare in Europa per affermare non solo quello che il settore agroalimentare ci richiede, ma anche quanto la scienza ha affermato e convalidato in tutti questi anni. La nostra dieta mediterranea deve essere valorizzata o i nostri prodotti di eccellenza, che ne fanno parte e tra i quali rientra anche il buon bicchiere di vino rosso, devono essere necessariamente valorizzati e non messi in un angolo, attraverso un meccanismo che poco ha di scientifico, perché non vede l'insieme l'insieme di una dieta e dello stile di vita di una persona, come fa la dieta mediterranea. Signor Ministro, lei deve portare in Europa la voce di una Nazione che ha sempre avuto un ruolo preminente

un insieme di principi e modelli, un paradigma etico-pratico che mette insieme tradizione, innovazioni, ecologia integrale e sviluppo sostenibile. È diventata patrimonio immateriale dell'UNESCO certamente perché si celebrano le proprietà salutistiche, ma anche perché portatrice di un immenso valore culturale ed è un vettore essenziale della qualità ambientale, sociale e culturale. Se tutto ciò è vero,

sulle etichette alimentari, perché lo scontro tra nutri-score francese e nutrinform battery italiano determinerà la dieta di milioni di persone e, di conseguenza, anche i costi che si riverseranno sul Sistema sanitario, se è vero che più ci si discosta dagli schemi della dieta mediterranea più aumentano le malattie cardiovascolari, e questo è scientificamente provato. Allora io dico: prendiamo il meglio dei francesi. Loro sanno comunicare molto bene attraverso l'informazione cromatica, che effettivamente arriva più facilmente al consumatore finale. Dobbiamo trovare quel punto di sintesi tra le informazioni puntuali e analitiche che noi fermamente fermamente sosteniamo del nutrinform con la cosiddetta capacità di portare al consumatore finale dette informazioni attraverso l'utilizzo di modelli cromatici.

quella griglia di informazioni che ampiamente sosteniamo proprio per dare contenuto scientifico alla qualità dei nostri alimenti. Questo è il mio suggerimento.

Signor Presidente, mi si consenta di fare un breve *excursus* per contestualizzare la nostra posizione dedotta nella mozione congiunta con i colleghi di Forza Italia. L'Italia, L'Italia, quando sin dal 1997 decise di introdurre la fece una scelta lungimirante, nella consapevolezza che dalla sicurezza alimentare deriva una sana popolazione. Ciò significa non solo longevità, ma minor spesa sanitaria. Altrettanto lungimirante fu quando nel 2003 si decise di portare a Parma l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonostante qualche recente svarione sulle fonti proteiche alternative, cui pensiamo si dovrebbe porre qualche rimedio. Ebbene, questi antefatti debbono metterci nella condizione di tenere fede in continuità alla *ratio* che li aveva ispirati, andando oltre la necessità di semplificare, assicurando al consumatore che il suo diritto all'informazione sia precipuamente finalizzato al suo benessere, conseguente a una più consapevole educazione alimentare e alla cultura dei sani stili di vita. Convinti che la tutela della salute umana e quella animale sono binomio inscindibile, e i virus pandemici ne sono la controprova, dovendosi superare l'indifferenza degli sprechi - e ve ne sono in sanità come in agricoltura - coniugando controlli, prevenzione, appropriatezza ed economia circolare. Da qui la centralità dei controlli nell'intera filiera agroalimentare per porre l'alimentazione quale primo gradino della prevenzione, a cominciare dal fatto che i sani alimenti sono l'architrave di un efficiente sistema immunitario. È per questo che, con il disegno di legge n. 1660, abbiamo inteso alzare ulteriormente l'asticella, con l'obiettivo di far emergere le criticità del nutri-score, investendo in prevenzione, controlli proattivi, sanità pubblica veterinaria, formazione specialistica innovativa, lotta all'antimicrobico-resistenza e valorizzazione delle produzioni di eccellenza, certi che nella sicurezza alimentare siamo *leader* europei e, come tali, dobbiamo comportarci e agire. Tutto questo è perfettamente in linea con le finalità delle altre mozioni presentate. n. 1660, infatti, non prevede solo di andare a recepire evolutivamente le normative europee, ma interviene per correggere le intrinseche incongruenze del nutri-score, valorizzando la dieta mediterranea con un sistema di valutazione secondo principi di trasparenza, tracciabilità e responsabilità, basato su indicatori ragionati e oggettivi, atti a qualificare le vere eccellenze della filiera, a garanzia dell'appropriatezza nutrizionale della giornata alimentare del consumatore. Un modello di *rating* dei prodotti agroalimentari replicabile su scala europea, perché siamo convinti che, solo assicurando una sana alimentazione, si può anzitutto migliorare la salute dei cittadini, coniugando e riqualificando la spesa sanitaria, con una strategia stringente di tutela dei consumatori riguardo alla composizione degli alimenti. sui cambiamenti nei modelli di consumo degli stessi, orientati a longevità e benessere, per far sì che l'allungamento dell'età media porti il consumatore in salute in età avanzata, contrastando le patologie tumorali derivanti dai determinanti ambientali *(Applausi)*, le patologie croniche,

che devono essere necessariamente fatte con materia prima territoriale, non importa se non in grado di soddisfare tutta la domanda mondiale, ma deve essere ben chiaro che deve trattarsi di prodotto alto di gamma, sostenuto dalle istituzioni con soli incentivi di comunicazione e d'immagine, posto che il prezzo deve essere tale da remunerare la qualità del prodotto. Per tutte queste ragioni riteniamo che, approvando la nostra mozione, ovvero nel contesto di un ordine del giorno che faccia sintesi di tutte quelle presentate, non ci possa essere migliore auspicio per il futuro della nostra filiera agroalimentare e per il ruolo guida che dobbiamo rivendicare, non solo nella sicurezza alimentare, ma anche nella prevenzione e promozione della salute, sostenere, con ampia partecipazione, l'approvazione del nostro disegno di legge legge n. 1660, nella revisione ordinamentale che deve accompagnare l'attuazione del PNRR.

l'attenzione e la cura per il prodotto italiano ci hanno contraddistinto da sempre, dal manifatturiero all'agroalimentare, tanto da occupare lo scenario mondiale nel mercato dei prodotti di qualità certificati ad indicazione geografica e biologica: tanti prodotti italiani, apprezzati a livello mondiale, a partire dai vini, dagli spumanti, dall'ortofrutta, dai salumi e dai formaggi, tutti di qualità. Questi prodotti si concretizzano nella cosiddetta dieta mediterranea. La dieta mediterranea è importante per tante ragioni. La dieta mediterranea è un patrimonio di conoscenze; è qualcosa che si è elaborata nei secoli e che tiene conto della stagionalità, della necessità di sostanze e degli apporti energetici che sono diversi a seconda delle stagioni. La nostra dieta mediterranea ha la caratteristica di essere equilibrata nei suoi principi. È varia e completa, dai grassi alle proteine. essa è - come tutte le diete - una sorta di lingua, di patrimonio identitario, che si è evoluta nel tempo. Gli elementi costitutivi della dieta mediterranea, come le melanzane, i pomodori, le patate, sono di origine straniera, americana, ma sono stati integrati e hanno trovato una loro armonia. Quindi, andare a estrapolare alcuni elementi, ad esempio l'olio, e valutarlo solo dal punto di vista dei grassi o degli zuccheri, non ci fa comprendere la sua completezza, che è tutto un insieme, è un ecosistema. La dieta mediterranea copre ogni stagionalità e, con un sapere secolare, tiene conto del fabbisogno degli apporti energetici diversi del nostro metabolismo, che varia durante dell'anno: nulla di più distante dal cibo standardizzato che ci propongono le multinazionali, che inganna con la chimica il nostro palato e, nel tempo, danneggia la nostra salute. salute. Entrando nel merito dell'oggetto della discussione sulla seguente mozione, risultano essere meritevoli di attenzione tre aspetti importanti: il primo, ovvero, i prodotti a base di vino dealcolato; il secondo il cibo del futuro e il terzo il nutri-score.

un sistema di etichettatura dei prodotti alimentari che fa emergere una classificazione dei valori nutrizionali. Iniziamo a chiarire il primo punto, ovvero i prodotti a base di vino dealcolato. Da un lato, si vuole colmare un vuoto normativo rispetto alla denominazione di vendita di alcuni prodotti; lato, vi è la valutazione se consentire il reintegro del volume perso in alcool, con acqua, nei vini dealcolizzati. Il Parlamento europeo si è già espresso negativamente per i vini a indicazione geografica (DOCG, DOC, IGT), lasciando comunque uno spiraglio sui vini da tavola. In Europa si sta tentando di rendere armonica una pratica che è già stata adottata in alcuni Paesi dell'Unione e proprio in questi giorni si sta dibattendo in Europa riguardo all'inserimento o no, via PAC, di questi prodotti all'interno del comparto del vino. In Italia il mondo vitivinicolo - da una parte - vede in ciò uno scandalo, in quanto si configurerebbe davvero come un annacquamento, ma - dall'altra parte - c'è invece chi intravede delle nuove opportunità. delle nuove opportunità. Il secondo aspetto riguarda i prodotti derivanti dalla forma larvale delle specie di insetti essiccati termicamente, di cui fanno parte sette specie autorizzate già nell'ambito dei mangimi per l'acquacoltura, ma per il *food* abbiamo soltanto il *tenebrio molitor* autorizzato dagli Stati membri Si tratta di prodotti già commercializzati in molti Stati membri e ovviamente ognuno fa capo alla propria legislazione nazionale. Con questo passaggio si intende armonizzare quella norma, per la loro commercializzazione, a garanzia del consumatore. Il terzo punto riguarda infine il nutri-score, ovvero il sistema di etichettatura a colori che danneggia la produzione *made in Italy* e soprattutto è asimmetrico informativamente nei confronti del consumatore. consumatore. Verosimilmente l'etichettatura nutri-score, come il modello francese, a semaforo, risulterebbe fuorviante per un'effettiva dieta bilanciata, con il rischio di penalizzare cibi salutari e promuovere cibi spazzatura. L'Italia su questo punto propone un'alternativa, ovvero il cosiddetto schema a batteria, per cui simili modelli non possono essere obbligatori e altresì non bisogna escludere l'applicazione obbligatoria per le produzioni a indicazione geografica, perché forme di espressione e presentazioni supplementari devono essere sostenute da elementi scientificamente fondati, per cui si dimostri che il consumatore medio possa comprenderne il reale e veritiero messaggio. Pertanto ritengo necessario che sia innescato tutto un sistema di prevenzione, tramite un'informazione adeguata ed etica, nell'interesse dei cittadini consumatori, che le nuove opportunità di mercato non compromettano i prodotti a denominazione di origine controllata, indicazione geografica tipica e denominazione di origine controllata e garantita per ciò che attiene i prodotti a base di vino dealcolato.

verso cui non dobbiamo avere nessun complesso di inferiorità. Così come con il nostro patrimonio rinascimentale abbiamo dato un contributo alla civiltà del nostro continente, allo stesso modo possiamo donare cibi salutari e un patrimonio alimentare di inestimabile valore, tornando alla dieta mediterranea, riconosciuta e apprezzata anche dall'UNESCO.

quello per cui il cibo in Italia non è soltanto un alimento o un nutriente, ma è anche cultura, tradizioni e distintività. La mia presenza oggi è legata al valore che il cibo ha per il nostro Paese, anche sotto il profilo economico e dell'attrattività turistica. tutelare questa distintività non può non essere un elemento centrale nelle politiche del Governo e credo che tutte le mozioni che oggi sono state presentate vadano esattamente in questa direzione, per la richiesta forte di tutela della distintività del cibo italiano. C'è un percorso che ritengo sia necessario scongiurare prima possibile, chiarendo immediatamente, a livello europeo e internazionale, la posizione del nostro Paese. Il percorso che porta il cibo a diventare una *commodity* e quindi a perdere la distintività, ci porta, passo dopo passo, verso la produzione di cibo sintetico. Credo che questa sia la cosa da scongiurare ed è il motivo per cui tutti insieme, in Europa, diremo chiaramente che questo percorso vedrà sempre la contrarietà del nostro Paese. C'è un legame stretto - si è detto in molti interventi della discussione generale - tra l'alimentazione e la salute, anche come elemento di prevenzione. E tale elemento rafforza la necessità di difendere le produzioni agroalimentari italiane, perché la dieta mediterranea - come diceva la senatrice Tiraboschi - è patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO, proprio perché porta con sé la capacità e la possibilità di prevenire molte patologie, incidendo anche sulla necessità di intervento del Sistema sanitario, altro aspetto economico non indifferente.

Il valore della dieta mediterranea è messo in discussione, in questo caso, da un sistema di etichettatura che non è informativo, ma è di condizionamento del mercato e ha come obiettivo condizionare il mercato e non dare informazioni reali ai cittadini e ai consumatori. Infatti, assegnare un colore al cibo è un modo certamente immediato di far percepire qualcosa al consumatore, ma è assolutamente slegato dal reale valore nutrizionale di quel prodotto. Anche in questo caso cito la senatrice Tiraboschi: è fondamentale cogliere quel valore comunicativo - il semaforo, nell'immaginario collettivo, è percepito immediatamente, grazie a Dio, altrimenti agli incroci faremmo un sacco di incidenti quella percezione immediata deve essere il frutto di un algoritmo che calcola, in modo reale, quale sia la portata nutrizionale legata alla porzione di cibo che viene quotidianamente o a pasto assunta dai consumatori. Paragonare l'olio d'oliva a una bevanda gasata e zuccherina o il parmigiano reggiano ad altre tipologie di cibo, non percependo che c'è una differenza nella quantità di prodotto che ciascuno di noi assume quotidianamente, genera, appunto, una distorsione che diventa condizionamento. Su questo punto è chiaro ed evidente il sostegno al nostro sistema di etichettatura, al nutrinform battery, che peraltro abbiamo notificato a novembre del 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, Dicastero

come la Grecia, Cipro e la Romania, altri Paesi dell'Unione europea si stanno accodando; soprattutto il dialogo è in corso con la Polonia, la Slovenia, la Croazia, la Spagna e, da ultimo, anche con il Ministro francese. Sono dialoghi proficui e credo che la soluzione che troveremo andrà in questa direzione. Vi sono, poi, altri elementi molto importanti nei testi delle mozioni, ma non voglio dilungarmi.

proteine animali, e quindi gli onnivori. Tuttavia, credo anche che sia giusto che il mercato in qualche modo porti al consumatore tutto il *range* di offerta alimentare,

la confusione comunicativa non agevoli il consumatore nella sua scelta alimentare.

riconosce il valore delle produzioni italiane. La nostra sfida è non solo continuare ad avere produzioni che hanno a che fare con l'artigianalità italiana anche in campo alimentare, anche portare prodotti di qualità, che non devono annacquarsi nella quantità, a scalare i mercati internazionali dove si crea valore aggiunto. E dobbiamo poi avere la capacità di distribuire tale valore aggiunto all'interno della filiera perché arrivi alla parte più debole, che è quella dei produttori.

fatto salvo il resto del testo; che il quarto impegno inizi con le parole: «a valutare le misure necessarie affinché», fatto salvo il resto dell'impegno. Al punto 5) l'*incipit* potrebbe essere il seguente: «a proseguire con le opportune iniziative presso le competenti sedi europee, al fine di contrastare l'adozione del del nutri-score*,* cosiddetto sistema semaforo, come sistema di etichettatura nutrizionale comune a livello europeo, suscettibile di veicolare», e fatto salvo il resto. Chiediamo poi di riformulare integralmente segue: «a studiare forme di incentivazione che consentano alle aziende che utilizzeranno il marchio nutrinform battery di coprire parzialmente le spese sostenute per l'adeguamento delle etichette.

primo impegno, che cito: «ad effettuare studi scientifici sulla valenza nutrizionale degli insetti che prevedano anche una valutazione di impatto sull'economia, sulla cultura alimentare e sui paesaggi e sulle tradizioni dei sistemi alimentari italiani ed europei» e con che cito: «a combattere lo spreco alimentare attraverso adeguate politiche che comprendano la promozione del recupero delle eccedenze alimentari, sia attraverso gli enti caritativi sia attraverso approfondimenti per lo sviluppo di piattaforme digitali che consentano di incentivare la pratica dell'utilizzo degli avanzi giornalieri nei supermercati e nei ristoranti».

Con la mozione oggi in discussione di Italia Viva-PSI siamo chiamati ad affrontare uno dei temi cruciali che coinvolgono il nostro Paese, quello della malnutrizione, e contestualmente parliamo di spreco alimentare. Le perdite e gli sprechi alimentari rappresentano una grande sfida per la nostra epoca, tanto più in un periodo in cui questo tema, purtroppo, si è dovuto affrontare in maniera molto più in maniera molto più incisiva a causa della pandemia. Dobbiamo trovare gli strumenti per debellare la piaga alimentare: circa 690 milioni di persone oggi soffrono la fame, mentre sono oltre tre miliardi coloro che non possono permettersi un'alimentazione sana. La pandemia non ha fatto altro che acuire il problema, mettendo a repentaglio la sicurezza alimentare e nutrizionale di un numero ancora più alto di persone. A questo quadro, che è drammatico, si devono aggiungere il deterioramento degli ecosistemi e l'impatto dovuti ai cambiamenti climatici. Parallelamente, le perdite e gli sprechi alimentari non accennano a diminuire

La discussione che questi numeri stimolano ci deve portare, quindi, a considerare la questione alimentare come una priorità. Proprio su questo profilo, l'Unione europea sta facendo dei passi avanti molto importanti, soprattutto con riferimento alla produzione di un nuovo tipo di alimento, basato sugli insetti, e pensato anche per far fronte a una graduale diminuzione di cibo, ovvero a un aumento di domanda dello stesso, in seguito ai cambiamenti climatici, alle carestie e alle pandemie di cui parlavo in precedenza. In questo senso, il piano d'azione dell'Unione europea 2020-2030 per i sistemi alimentari sostenibili identifica proprio gli insetti come una fonte di proteine a basso impatto ambientale, che può sostenere la transizione verde della produzione alimentare dell'Unione europea stessa. Gli Stati membri hanno autorizzato recentemente la commercializzazione delle cosiddette tarme della farina, che potranno quindi essere immesse in commercio come farina, prestandosi adesso in un ingrediente fondamentale per numerosi prodotti alimentari. È il primo assenso dell'Unione europea ad un insetto come alimento, che arriva a seguito della valutazione scientifica da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Per l'Europa, ovviamente, gli insetti sono un cibo nuovo, estraneo alla cultura popolare, anche se in alcune culture vengono consumati da molto tempo. A regolarne l'ingresso sul mercato interno dell'Unione europea è il regolamento sui nuovi prodotti alimentari del 15 maggio 1997: il regolamento prevede ovviamente una valutazione stringente, condotta dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che deve concludere che quel cibo non comporta rischi per la salute umana. Chi vi parla è sardo e in Sardegna è noto che il cosiddetto formaggio marcio, che tutti conoscono per la presenza di vermini piccolissimi, è un alimento estremamente diffuso con un potere nutrizionale elevatissimo, che adesso inizia ad ottenere il riconoscimento anche da parte degli organi preposti. Fino a poco tempo fa era addirittura vietato, ma da sempre costituisce un cibo fondamentale, molto rinomato e ricercato in Sardegna. Le larve della tarma della farina di cui prima ho parlato - sono i primi insetti autorizzati come cibo, ma non saranno sicuramente gli ultimi, visto che ci sono undici richieste per insetti da utilizzare come cibo al vaglio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Secondo la FAO, l'uso degli insetti come alimento per l'uomo diviene particolarmente rilevante a causa del costo crescente delle proteine animali, dell'insicurezza alimentare, della crescita demografica e della crescente domanda di proteine da parte delle classi medie ed è sicuramente necessario trovare soluzioni alternative all'allevamento convenzionale. Il consumo di insetti contribuirà quindi positivamente alla tutela dell'ambiente e della salute.

Si tratta quindi di cibi che possono essere coltivati e allevati in sistemi modulari, che riducono l'esposizione a rischi ambientali e non richiedono neanche troppo consumo di suolo. Sarebbero quindi adatti anche ad ambienti urbani, oppure ad isole magari distanti dalla terraferma.

l'utilizzo di insetti per risolvere alcune problematiche alimentari non costituisce in alcun modo un attacco alla dieta mediterranea. L'utilizzo di proteine nobili degli insetti infatti è molto diffuso in altri Paesi, ma appare incapace ma appare incapace di sostituirsi alle proteine nobili appartenenti alla nostra cultura gastronomica. Si tratta quindi di proteine destinate in maniera settoriale solo ad alcuni comparti alimentari e nulla avrebbero a che fare con le proteine della dieta *made in Italy*. Quello che invece siamo chiamati a fare è cogliere gli aspetti più positivi, quelli che ci consegnano un'opportunità imprenditoriale, anche se resta, ferma e salda, la difesa delle produzioni tradizionali che caratterizzano il nostro *made in Italy* e la dieta mediterranea. Peraltro, proprio la trasformazione ecologica rappresenta il 40 per cento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, consentendo ai nuovi operatori e sistemi produttivi di creare nuovi posti di lavoro. Dobbiamo quindi incentivare queste diverse possibilità, seppure nel pieno rispetto della conoscibilità e dell'informazione da parte dei consumatori finali circa la natura di nuovi prodotti alimentari che saranno immessi nel commercio. Auspico quindi che la mozione che abbiamo presentato come Italia Viva-Partito Socialista Italiano, possa fungere da stimolo e da impegno per il Governo per incrementare lo studio di proteine alternative, come quelle degli insetti, avendo cura di contemperare esigenze diverse, ma tutte meritevoli di tutela; da un lato, l'esigenza rappresentata dall'industria e dall'imprenditoria, dall'altro, la salvaguardia della nostra tradizione, facendo chiarezza sui metodi di produzione e sulla stessa provenienza del cibo, considerato anche che la maggior parte dei nuovi prodotti proviene da Paesi extraeuropei. Al contempo è necessario avviare ogni utile iniziativa per combattere lo spreco alimentare sia attraverso campagne di sensibilizzazione, sia tramite lo sviluppo di piattaforme digitali, che consentano di incentivare la pratica dell'utilizzo degli avanzi giornalieri nei supermercati e nei ristoranti, altro tema di estrema rilevanza. Occorre rivolgersi direttamente all'intera comunità affinché ci si impegni a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari e al recupero quindi di quel tipo di cibo, così da evitare un ulteriore tracollo della sicurezza alimentare e un impoverimento delle risorse naturali.

ed è anche un ottimo segnale. Come non è un caso che ancora una volta sia Fratelli d'Italia a sollecitare il dibattito parlamentare sul tema della difesa dei prodotti e dei produttori italiani. Non è un caso perché, come abbiamo sempre detto, il nostro unico interesse era, è e sarà sempre l'interesse nazionale. Non è un caso nemmeno perché lo abbiamo detto sin da subito che saremmo stati utili, anche senza entrare in questo Governo; un Governo più di grandi compromessi che di larghe intese. Saremmo stati utili e lo siamo, senza chiedere nulla in cambio. Siamo utili oggi più che mai per sollecitare l'intero Parlamento a porsi come argine ad una deriva verso la quale questa Europa, sempre sempre più della finanza e sempre meno dei popoli e delle Nazioni, sembra inesorabilmente destinata. Un'Europa che calpesta le sue stesse radici, la sua cultura, le sue tradizioni e i suoi millenari saperi, in nome di un ordine nuovo nuovo che ci vorrebbe tutti ridotti a meri consumatori con gli stessi gusti ed orientamenti, facilmente addomesticabili e quindi facilmente governabili. Insomma qualcosa di lontano anni luce dall'idea di libertà, ma anche dall'idea stessa di Europa. Lasciare che siano gli interessi di pochi a condizionare la vita dei popoli non è lo spirito con cui abbiamo a fatica costruito la civiltà in cui abbiamo la fortuna di essere nati e che abbiamo il dovere di rispettare e perpetrare. È proprio per combattere questa visione che Fratelli d'Italia ha chiesto di discutere una mozione per tutelare le nostre tradizioni, i nostri saperi e le nostre genti. Come l'anno scorso a febbraio avevamo fatto alla Camera e come anche quest'anno abbiamo fatto - Ministro, lei lo sa - in un *question time* incentrato proprio sul nutri-score. una mozione che impegna tutto il Senato ed il Governo a dire no a chi vuole chiamare vino una bevanda che vino non è, a dire no a chi vorrebbe chiamare carne una poltiglia vegetale o peggio ancora un artefatto sintetico, a dire no a chi vorrebbe sostituire la dieta mediterranea - che ricordo è patrimonio UNESCO - con cavallette, larve ed altre amenità fritte, a chi vorrebbe con i nutri-score discriminare i prodotti tradizionali per far spazio a quelli costruiti in laboratorio in nome di una presunta salubrità tutta da dimostrare, anzi indimostrabile perché assolutamente scorretta, e infine a dire no a chi vorrebbe penalizzare ancora i nostri prodotti con l'*italian sounding.* Fugo subito ogni dubbio sul fatto che vogliamo in qualche modo censurare o limitare le libertà di chi sceglie di cibarsi di larve ed insetti: per noi chiunque può sentirsi libero di mangiare ciò che più gli aggrada, sia chiaro. Quello che non vogliamo è la demonizzazione dei nostri prodotti tradizionali, per cui mangiate pure cavallette e larve, ma non diteci che sono migliori dei nostri prodotti tradizionali. Per evitare che ciò accada, oggi non basta più una semplice enunciazione di principio, ma serve una presa di coscienza scevra da condizionamenti ideologici che portano qualcuno ad occuparsi di cambiare la Costituzione, sentendosi magari al pari dei Padri fondatori senza aver preso però nemmeno un voto alle elezioni del proprio condominio, per inserirci la tutela ambientale e girarsi invece dall'altra parte quando quelli che l'ambiente lo difendono da sempre si vedono sotto costante attacco. Sì, perché quelli che da sempre giocano un ruolo fondamentale nella gestione dell'ambiente sono gli agricoltori, che lo fanno dalla notte dei tempi, mentre chi oggi si riempie la bocca di sostenibilità fino a ieri, ma forse anche oggi che ne parla, non ha mai pulito un sentiero, coltivato un orto o munto una vacca. demagogia, non è una banalità come quelle che sento spesso in quest'Aula quando si parla di ambiente, ma è l'essenza stessa dell'approccio che noi conservatori abbiamo nei confronti dell'ambiente. Ci siamo sempre occupati della nostra terra, della nostra Patria, convinti come siamo che la cura dell'ambiente passi attraverso la cura di quello che sentiamo nostro, di quello che sentiamo vicino, di quello che noi chiamiamo casa o Patria. Anche oggi vi invitiamo ad occuparvi quindi dei problemi concreti e reali che i nostri produttori, spesso da soli, affrontano per fare in modo che in tutto il mondo si possano apprezzare i nostri prodotti, perché non potrà sfuggirvi che siamo sotto attacco e che dobbiamo difenderci adesso tutti e senza indugi. un'opposizione patriottica e soprattutto responsabile, non segnaliamo mai un problema senza dare una soluzione, consci come siamo che segnalare un problema senza dare una soluzione ci fa diventare parte stessa del problema. Noi non vogliamo essere un problema, ma saremo di qui a poco la soluzione del problema di questa Nazione. Oggi però, con lo stesso spirito responsabile, vi diciamo quanto sommessamente crediamo possa essere utile, quello che fuori di qui la gente sa essere utile, soprattutto quei produttori che, contrariamente a chi si crede

più esperte del sistema, possano provare l'inutilità scientifica del sistema nutri-score e che anzi aiutino e sostengano quello che il Ministero ed il Ministro hanno già fatto attraverso il decreto per l'introduzione e la sperimentazione del nutrinform. questa sperimentazione, che deve passare per forza attraverso i dati raccolti dalle aziende, non sia a carico dei produttori, altrimenti ci ritroveremo cornuti e mazziati, ma che tutto o parte di quel costo o parte di quel costo venga sostenuto dallo Stato, consci dell'importanza che quei dati avranno in sede europea quando dovremo dimostrare l'efficacia del nutrinform rispetto al nutri-score.

del *farm to fork,* di cercare un'etichetta armonizzata. Dobbiamo fare fronte comune con quelle Nazioni che hanno capito l'inganno che c'è dietro, a quelle Nazioni che non si fanno certo abbindolare dalle multinazionali, dalla finanza e dalle sponsorizzazioni, ma che credono invece che la vera forza dell'Europa sia la diversità, la sua biodiversità, ma anche il suo diversismo. Noi siamo diversisti da sempre, siamo contro l'appiattimento, siamo contro la globalizzazione, non abbiamo mai vissuto in paradisi dove tutti erano uguali e tutti al ribasso come nei paradisi comunisti, non li abbiamo mai idolatrati come gran parte di questo Parlamento, quindi siamo forti della nostra cultura che regaliamo

del clima sono carne sintetica e insetti. Questo non è il mondo in cui vogliamo vivere; questa non è l'Europa dei popoli che abbiamo contribuito a costruire; questo non è il mondo che vogliamo lasciare ai nostri figli.

un'idea complessiva di qualità che vogliamo fornire al consumatore attraverso i nostri prodotti. Questo radicato modo di concepire il rapporto con gli alimenti e l'alimentazione è un patrimonio

dire per pochi altri posti nel globo) un radicamento profondo nella storia, nelle tradizioni e nella cultura, di cui sono in qualche misura l'espressione trasmessa dalle generazioni nel tempo. Credo che

e anche dei consumatori, che hanno il diritto di avere tutte le informazioni e gli elementi per poter scegliere e decidere cosa utilizzare nella loro vita. Credo anche di poter dire che questa concezione di agricoltura, alimentazione, cucina e tradizioni sia all'origine della percezione, che presenta a livello globale, di un un mondo da cui provengono cibi autentici e di qualità. Credo che gran parte di quell'immagine del *made in Italy* come luogo di produzione di autenticità e qualità abbia radici profonde in tutto questo.

Tra le questioni fasulle vorrei inserirne due apparse sui giornali nei giorni passati. La prima è quella legata agli insetti.

L'EFSA ha fornito un suo parere, sul quale un comitato tecnico della Commissione europea si è espresso favorevolmente. La questione riguarda l'armonizzazione delle normative a livello europeo.

Si è aperta una riflessione a livello europeo su quali siano le condizioni minime per cui poter ancora chiamare vino un prodotto che ha subito una drastica riduzione di alcol. Credo che questi siano temi da affrontare assolutamente nel merito perché qui, da una parte, è in gioco l'idea e la tutela dell'identità di un prodotto come il vino che è caratterizzante per i nostri territori, la nostra cultura e le nostre tradizioni. Dall'altra parte, occorre fare una riflessione molto seria e pacata

mozione - che il Ministero debba muoversi su questo tema con grandissima attenzione, perché va fatto tutto il possibile per rispondere ai bisogni reali, ma avendo ben chiaro che non si deve intaccare la nostra idea

uno scontro culturale in atto tra un'idea di agricoltura come la nostra, rispettosa del legame con i territori, le tradizioni, le culture, la storia, la trasparenza e l'autenticità dei prodotti

tra l'altro sventagliando alcune questioni che hanno una presa. Quando parliamo infatti di dare informazioni semplici e facilmente comprensibili al consumatore,

È chiaro però che se la scelta per fare questo è definire un colore di semaforo sulla base delle calorie, degli zuccheri o dei sali presenti in 100 grammi di prodotto, comparando un bicchiere d'acqua minerale con un vino stagionato di grande qualità, questo ragionamento non sta in piedi e non è percorribile. Bisogna fare attenzione perché questo è uno dei temi in gioco. C'è poi tutta la questione di non fornire indicazioni che ledano la concorrenza:

esiste il tema dell'*italian sounding*, perché la percezione globale dei nostri prodotti è talmente alta che molti cercano di speculare provando a emularla. Non per nulla esiste un riconoscimento importantissimo della dieta mediterranea da parte dell'UNESCO,

mozioni dia forza al Ministro per farlo. Credo che il tema sia anche quello delle alleanze. Questa partita, al di là delle buone intenzioni, la vinceremo se sapremo fare blocco, a livello europeo, con tutti coloro che cominciano a capire che il nostro punto di vista è importante per il Paese. Voteremo a favore di queste mozioni proprio per dare forza al Ministro e per portare la nostra idea di rispetto dei consumatori e della qualità degli alimenti in Europa e nel mondo.

il nostro Paese, proprio nel campo dell'agroalimentare e dell'agricoltura, ha fatto dei passi in avanti giganteschi.

non si sono succedute da un Governo all'altro, ma hanno avuto un tratto distintivo molto chiaro. Tali scelte hanno puntato, quasi esclusivamente, sulla qualità e sulla distintività dei nostri prodotti agricoli e della nostra agricoltura. Anzi, vorrei dire qui delle nostre agricolture, perché la vera forza dell'agricoltura italiana è il fatto che di tante agricolture. C'è l'agricoltura di montagna e quella legata ai territori; è il tratto della distintività della territorialità.

vi è stato uno sforzo gigantesco, che, puntando sempre di più sulla qualità, sulla ricerca legata al territorio, sulla distintività dei prodotti, ha conquistato tutti i mercati internazionali, facendo sì che proprio il campo dei prodotti a denominazione di origine diventasse la nostra punta di diamante. È diventato anche un approccio culturale molto forte. Vorrei ricordare che una delle leggi che ha rappresentato in qualche modo una svolta

negli ultimi cento anni, anche nel nostro Paese, si è perso un numero enorme di specie e di semi. Quindi, quella legge ha rimesso in movimento tutto il settore e ha fatto sì che ci fosse

è una sorta di risposta, dall'altra parte, a questa nostra battaglia, che non è solo sull'etichettatura, ma anche sull'origine dei prodotti, che dà forza ai territori che li producono e agli agricoltori.

iniziative e sul lavoro e, quindi, vanno bene le mozioni e dobbiamo ricordare che, purtroppo, vi è una penalizzazione anche in alcuni trattati commerciali. So che a molti non farà piacere che lo cito, ma vi sono alcuni trattati commerciali che non ci aiutano a valorizzare i nostri prodotti agroalimentari e che rischiano di essere dannosi. Credo quindi che, nel portare avanti e sostenere

andiamo a firmare alcuni trattati commerciali. Cito il CETA, ma potrei citarne qualcun altro. In Europa l'iniziativa per fermare operazioni come quella del nutri-score si

le mozioni che ci apprestiamo a votare sono fondamentali per fare chiarezza e ribadire l'impegno di questa maggioranza a sostegno delle eccellenze agroalimentari italiane: un settore che vale ben 500 miliardi. Per avere contezza, vale precisamente ben il doppio del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Paragono le due cose perché, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza l'Europa ci ha teso una grande mano per la ripartenza, e di ciò dobbiamo essere grati. Sono una convinta sostenitrice dei valori europei; lo è anche il Gruppo a cui appartengo e di cui oggi sono voce: Forza Italia. Allo stesso tempo, però, quando le cose non vanno bene, dobbiamo far comprendere che la strada intrapresa evidentemente non è quella più giusta ed equa da percorrere. Forza Italia, sia nel Parlamento europeo che in Italia, è da sempre schierata contro il sistema del nutri-score; lo abbiamo sempre ribadito a gran voce senza indugi. Credo che la chiarezza sia un punto di partenza imprescindibile, così come imprescindibile e costante deve essere l'impegno a tutela dell'unico settore che ha resistito allo tsunami della pandemia. Quando molte attività erano chiuse, quando i container a transitare da una parte all'altra del mondo erano davvero pochi, il *made in Italy* continuava a correre veloce, espandendosi in mercati nuovi, come ad esempio l'*e-commerce*. Solo in Italia, nel 2020, l'acquisto di generi alimentari ha raggiunto i 2,5 miliardi, registrando un più 55 per cento. Nel mondo si stima che un consumatore su dieci consumi cibo italiano. Quello delle esportazioni è un settore che vale 46 miliardi; non è prevista alcuna flessione. L'agroalimentare è una vera e propria certezza per il nostro PIL, così come l'estensione del *golden power* dimostra: c'è necessità di estrema attenzione e netto contrasto perché il nutri-score non è solo un nodo da sciogliere prima dell'accordo sulla nuova PAC. Esso costituisce piuttosto un vero e proprio attacco alle nostre eccellenze, alla nostra qualità. È chiaro che la politica europea - secondo le ultime decisioni - mira tra l'altro a sostenere scelte alimentari basate su prodotti vegetali. Sono ormai esplicite le aperture ai sostituti di carne e formaggi, hamburger e bistecche vegane, farine di tarme come cibo sostenibile. Al riguardo vorrei ribadire quello che ho già espresso martedì in Aula. In Italia il comparto agricolo, custode delle nostre magnifiche terre che ci regalano cibo di qualità, ha fatto passi da gigante in materia di sostenibilità ambientale, prima ancora dell'arrivo della batteria di aiuti a sostegno della sostenibilità e dell'economia circolare. In materia agricola siamo il Paese più *green* d'Europa, questo primato lo dobbiamo proprio all'impegno dei nostri agricoltori a tutela della biodiversità, alla diffusione del biologico, all'efficienza nell'uso della chimica e dell'acqua. Al riguardo ricordiamo il taglio pari al 20 per cento dell'uso dei pesticidi tra il 2011 e il 2018, al contrario della Francia, della Germania, dell'Austria, dove l'utilizzo dei prodotti fitosanitari è addirittura aumentato del 39 È quindi evidente come la nostra agricoltura riesca a coniugare in maniera efficiente tutela dell'ambiente e qualità delle produzioni, contribuendo in maniera determinante alla crescita economica del Paese. Al Governo si chiede quindi di promuovere maggiormente in Europa questa realtà *green* italiana. Anche così, ne sono certa, la dieta mediterranea vincerà sull'idea di un'alimentazione che invita, noi e i nostri figli, a consumare menù a base di latte di piselli, di hamburger vegetali, di tarme di farina e, per mandare giù il boccone, del vino dealcolizzato. È quanto mai necessario approfondire, con specifici studi scientifici, questi cibi alternativi, per dare dati certi su valori nutrizionali e impatti culturali. I tre miliardi che l'Europa pensa di investire da qui al prossimo futuro per la promozione dei cibi alternativi potrebbero essere, ad esempio, usati anche per avviare campagne informative su regimi alimentari equilibrati e allo stesso tempo bio, con i tipici elementi che da sempre accomunano la cultura culinaria italiana ed europea. Dico ciò perché non siamo solo noi di Forza Italia a rimanere basiti di fronte ad alcune ricette sostenibilmente alternative, lo sono soprattutto gli italiani che, per la maggior parte, considerano cibi come ad esempio gli insetti estranei alla nostra cultura alimentare. Quali sarebbero, poi, gli *standard* di sicurezza alimentare? Me lo chiedo perché noi italiani imprenditori del settore siamo molto scrupolosi al riguardo. Investiamo oltre 3 miliardi l'anno per garantire sicurezza e qualità ai nostri prodotti. Riguardo ai prodotti alternativi ci aspettiamo, quindi, rigorosi controlli. Questi sono i motivi per cui noi di Forza Italia chiediamo il massimo impegno nel creare un fronte comune in Europa contro l'adozione di pratiche come l'etichetta semaforo, inaccettabile per il nostro Paese e le nostre produzioni. Con questa etichetta, le eccellenze delle nostre tavole finirebbero per perdere *appeal* rispetto ai prodotti come la Coca-Cola, che avrebbero semaforo verde a discapito, ad esempio, al nostro olio di oliva, contrassegnato purtroppo con il rosso. Si perderebbe, in questo modo, anche la centralità delle indicazioni in etichetta dei valori nutrizionali, che verrebbero privati della loro importanza. L'equiparazione verrebbe fatta solo prediligendo un prodotto con un costo inferiore e sappiamo bene che gli elementi italiani hanno un prezzo elevato perché il costo di produzione è maggiore, proprio in virtù dei nostri elevati *standard* qualitativi. Chi acquista italiano acquista prima di tutto qualità e questo possiamo ribadirlo con fierezza. chiedo un impegno deciso sul contrasto alla concorrenza sleale in materia di costi produttivi, nonché del contrasto del fenomeno all'*italian sounding*, che, unito a quello della vera e propria contraffazione, è stimabile in 100 miliardi di euro a livello globale. In Europa, per esempio, sono molto imitati i sughi delle tipiche ricette italiane i quali costituiscono il 55 per cento del fenomeno dell'*italian sounding* nel vecchio continente. continente. In conclusione, sì, bisogna omogeneizzare sicuramente il sistema di etichettatura europeo, ma bisogna farlo nella maniera più completa, imparziale e rispettosa possibile. Ecco perché, noi di Forza Italia, promuoviamo da sempre il nutrinform battery, il sistema a batteria. Lo facciamo anche oggi, in questa mozione, insieme ai colleghi della Lega. Per questo motivo, che si aggiunge agli altri già elencati, annuncio naturalmente il voto favorevole del Gruppo Forza Italia e ringrazio il Ministro per la chiarezza con la quale oggi in quest'Aula ha ribadito come sia necessario rispondere alla richiesta pervenuta da tutti sulla tutela della distintività nazionale. Sono certa che la battaglia sul nutri-score ci vedrà vincitori insieme ai 313 prodotti con marchio di qualità che sono delle vere e proprie medaglie al valore per il nostro *made in Italy*.

abbiamo già detto più volte, la filiera del cibo, compresa la ristorazione, il canale Horeca e tutto il resto che rientra nella distribuzione e nella vendita, valgono oltre 520 miliardi. Rappresentiamo oltre il 25 per cento del prodotto interno lordo.

nel mondo? I conti sono presto fatti. 140 miliardi è il valore della nostra produzione ed esportiamo per 46 miliardi, nonostante la pandemia. L'*italian sounding*, le imitazioni del cibo italiano nel mondo, valgono 100 miliardi. Abbiamo anche la falsificazione vera e propria, che vale 60 miliardi per un totale di oltre 340 miliardi. È questo il valore vero del prodotto italiano nel mondo, se riuscissimo a coprire anche l'*italian sounding* e la falsificazione. Sono oltre 6.000 i diversi tipi di salumi, 430 i tipi di formaggio, 350 i tipi di salami, pani, uve e vino. Le DOP e le IGP, insieme ai vini, sono oltre 40 per ogni Regione italiana. Parliamo di oltre 5.000 ricette che alimentano la nostra cucina, con *standard* di qualità troppo elevati, al punto da innescare la pericolosa idea di eliminare o limitare la fastidiosa presenza dei prodotti alimentari italiani nel mondo. mondo. È in atto un attacco frontale, senza vergogna, al nostro stile alimentare e alla nostra dieta, che si basa sulla tutela dell'ambiente, sull'etica, sulla salute e sulla condivisione a tavola. *(Applausi)*. Sono temi importantissimi! Vediamo uno spettacolo vergognoso: partiamo dall'ONU, che prima ha dichiarato la nostra dieta mediterranea patrimonio mondiale dell'umanità e poi si contraddice nell'affermare che fa male, perché troppo proteica. Ci sono i gruppi multinazionali e le potenze economiche dietro tutto questo, perché consapevoli che oggi più che mai, nel mondo, chi è padrone della fame sarà il padrone vero del mondo. Molti dicono che la prossima guerra sarà per l'acqua, per il petrolio

capacità di interpretare questi segnali. Anche il prezzo dei piselli da proteina è alle stelle e cresce il mercato degli oli vegetali: sono segnali importanti, per far capire che sta cambiando la tendenza.

Tale commissione dispone di risorse economiche straordinarie ed intende proporre stili alimentari lontani dal nostro modello di dieta mediterranea, basati solo su studi epidemiologici, senza avere alla base nessun fondamento clinico che ne certifichi l'efficacia e la salubrità. Questo modello risulta avere delle gravissime carenze. Questi piani sono gravemente lesivi della libertà di scelta del consumatore, vorrebbero prevedere una guida delle scelte, attraverso incentivi e disincentivi a consumare un determinato tipo di prodotto e perciò un determinato tipo di dieta.

con 208 milioni di pezzi venduti. Rispetto agli ultimi due anni precedenti il mercato è già cresciuto del 38 per cento. Questa tendenza è contro il *made in Italy*: non dimentichiamolo mai. Tutto questo vuole condizionare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sull'assegnazione delle nuove risorse della PAC, mettendo dentro tutto quello che non è mai esistito nella tradizione contadina e nell'agricoltura del nostro Paese e che non fa parte della dieta mediterranea. pensar male su ciò che sta dietro questo attacco. L'Unione europea, con la presidente Ursula von der Leyen, per come si sta comportando non è assolutamente una sostenitrice del *made in Italy* anzi il suo credo è il nutri-score, che come abbiamo detto tutti prima - il Ministro non lo ha accennato, ma diciamolo chiaramente - premia la Coca-cola *light* rispetto all'olio extravergine di oliva. Ci sono poi, a livello mondiale, delle figure sponsorizzate da multinazionali, che fanno un po' da traino e da *leader* su questo aspetto. Sono le stesse multinazionali che fatturano decine di miliardi di euro con il cibo

Per ovvie considerazioni non cito i nomi di queste multinazionali, però è gravissimo. Pensate che, nel postare il video di latte a base di piselli, hanno avuto il coraggio di brindare, di dire «Salute!» e questo è assolutamente grave, non è ammissibile. Per non parlare, poi, dell'hamburger vegano, altro tema straordinario: 52 per cento di proteine di soia, 19 per cento di acqua e altre proteine di soia, oli vegetali, aceto, aromi. Ma questo è un hamburger, questo è il futuro? Per noi questo non è un hamburger e non è il futuro. La Commissione europea ha dato il via libera all'uso alimentare dei vermi, il *tenebrio molitor*; gli insetti fanno parte della strategia *from farm to fork* per la sostenibilità dell'alimentazione europea, con motivazione incomprensibile. La sostenibilità alimentare europea, da qui al 2030, dovrebbe aver dettato, sulla linea delle proteine, la valorizzazione degli insetti rispetto al resto, rispetto a quello che c'è già. Noi su questo siamo profondamente contrari. È necessario tutelare con determinazione le eccellenze alimentari italiane. Contraffazione, applicazione di misure protezionistiche, etichettatura ingannevole e fuorviante sono evidenze di un costante attacco all'agroalimentare italiano.

Ma noi, con il disegno di legge presentato dal Gruppo Lega, a prima firma della senatrice Cantù, AS 1660, vogliamo incentivare il raggiungimento di *standard* qualitativi elevati dei prodotti agroalimentari italiani, introducendo un sistema di *rating* per la certificazione di eccellenza, la riforma del sistema di prevenzione, la programmazione e il controllo vero della sanità pubblica.

dal punto di vista degli allevamenti intensivi, la zootecnia, siamo ad emissioni più basse rispetto a tutto il sistema europeo. Pertanto, sostenibilità, capacità di trasformare il benessere animale in attenzione particolare da parte dell'agricoltore e dell'allevatore, forza di volontà di andare incontro alle esigenze del consumatore finale, che - lo ricordo - è il datore di lavoro di tutta la filiera: non dimentichiamocelo mai, è fondamentale questo passaggio. Noi oggi vogliamo impegnare il Governo a una opportuna iniziativa, affinché venga accolta a livello europeo una posizione che coincida con la necessità di tutelare le denominazioni. Vogliamo che l'Esecutivo si attivi per la promozione del *made in Italy,* per il sostegno alle nostre aziende e alla filiera agroalimentare italiana, con ritorno, come si diceva in precedenza, alla prima parte della filiera.

signor Presidente, ricordo che dal tentativo dell'ONU di tre anni or sono, il nutri-score, oggi dell'Europa, fino all'ultimo attacco alla dieta mediterranea, questi attacchi nulla hanno a che fare con gli interessi che...

Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, colleghi, oggi siamo qui a sottolineare che le eccellenze delle nostre produzioni agroalimentari sono il frutto di secoli in cui c'è stata la massima integrazione tra tradizione e innovazione, tra il sapiente discernere tra ciò che è bene conservare e quanto è giusto innovare. La conformazione geografica del nostro territorio ci consente coltivazioni variegate e di qualità che, con l'abilità dei nostri produttori, hanno generato questo consolidato apprezzamento, diffuso in ogni parte del mondo. I numeri di questo prestigio internazionale sono racchiusi nelle produzioni certificate di qualità in costante crescita e nelle varie produzioni sempre alla ricerca del meglio. L'Italia primeggia nel mondo per la grande cura rivolta ai metodi di lavorazione del prodotto e alla trasparenza delle indicazioni in etichetta per fornire ogni possibile informazione atta a far compiere al consumatore una scelta più consapevole. Importante è la consapevolezza negli acquisti nella prospettiva di perseguire comportamenti salutari. Noi siamo ciò che mangiamo, quindi un risparmio a livello

sia tra i nostri consumatori che tra i nostri produttori. Si assiste a tentativi di offuscare il *made in Italy* attraverso improbabili soluzioni che avrebbero a che fare con la salute o la migliore commercializzazione del prodotto, ma che in realtà sembrano solo voler destabilizzare questa nostra supremazia nell'agroalimentare, a vantaggio di altri interessi particolari. prima fra tutti, all'etichettatura con il sistema nutri-score che, semplicistica e fuorviante, presenta elementi di contrasto con la bilanciata alimentazione della dieta mediterranea. Da questa indicazione, ad esempio, emerge il dato assurdo che l'olio di oliva non risulta tra gli alimenti consigliati, quando invece ci sarà un motivo se, dopo il latte materno, è il primo elemento inserito nello svezzamento del bambino. quindi, non è informativo, ma di condizionamento del mercato. Giustamente, sia in Parlamento che nel Governo, la posizione pressoché unanime è di contrasto a tale etichettatura. Ad ora, la proposta alternativa è la grafica informativa a batteria del nutrinform, pensata per fornire informazioni sull'apporto nutrizionale in rapporto al corretto stile alimentare, evidenziando la percentuale in calorie, zuccheri e sale presenti nel prodotto, senza stabilire a priori ciò che è assolutamente negativo da quello che è incontrovertibilmente buono. All'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è affidato il compito di fornire una consulenza scientifica sulle sostanze nutritive importanti per la salute pubblica, al fine di definire la strada da intraprendere per un'eventuale etichettatura univoca in Europa. Il parere dell'EFSA sarà rilasciato entro marzo del 2022, ma già entro la fine di quest'anno sarà indetta una consultazione pubblica sulla bozza. altro allarme è scattato alla paventata possibilità di abbassare il contenuto di alcol in alcuni vini, che ha subito trovato opposizione nello stesso Parlamento europeo, almeno per i vini a denominazione controllata. Le bevande dealcolate devono essere considerate come una categoria a parte e ben venga un prodotto alternativo, ma è bene sottolineare che in nessun caso può essere confuso con il vino, tanto più se viene considerata pratica enologica l'aggiunta di acqua. fermi tutti i limiti previsti dai disciplinari di produzione del vino, che hanno da sempre svolto la funzione di frenare queste derive qualitative. Attenzione doverosa deve essere posta anche all'armonizzazione normativa tra i Paesi membri circa il cosiddetto cibo del futuro, quello che fa riferimento alla farina gialla, ossia derivata dalle larve della specie di insetti *tenebrio molitor* essiccati termicamente,

Il periodo pandemico che stiamo vivendo ha evidenziato come il comparto primario sia ancora oggi, nell'era tecnologica, un settore vitale per l'umanità, che ha bisogno di produzioni sane e alla portata di tutti, in cui la trasparenza deve essere un impegno nella produzione quanto nella commercializzazione. In tale direzione vanno le scelte a livello comunitario del *green deal*, in cui la strategia dal produttore al consumatore trova ampio spazio e condivisione. Il MoVimento 5 Stelle da sempre si è impegnato a mettere in atto numerosi interventi per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari italiane nel mondo ed il contrasto alla contraffazione. L'*italian sounding* vale 100 miliardi, con un aumento *record* del 70 per cento nel corso dell'ultimo decennio, ed è una concreta minaccia alle cose buone che sappiamo fare e al nostro made in Italy. Il nome di un prodotto, unito alla propaganda commerciale, influisce non poco sui consumi e la standardizzazione di prodotti e sistemi produttivi di massa creano vantaggi alle grandi multinazionali, a discapito della varietà alimentare, delle piccole produzioni locali e delle tipicità a chilometro zero. Con questa mozione chiediamo al Governo di perseguire la massima trasparenza e corretta informazione a tutela del sapere e del fare tipico italiano; di proteggere la nostra produzione vitivinicola e favorire la diffusione di dati chiari e corretti sugli aspetti nutrizionali degli alimenti; di perseguire ad ogni livello politiche di sostegno alle nostre produzioni agroalimentari; di rafforzare il contrasto alle contraffazioni alimentari e sostenere la corretta educazione alimentare, basata sulla dieta mediterranea, che vede da sempre l'Italia protagonista e ora più che mai attenta all'incremento della biodiversità e alla tutela del lavoro agricolo. Per tutti questi motivi il MoVimento 5 Stelle ha lavorato

abbiamo fatto un bel dibattito importante, ma vi sollecito su un altro punto di vista. Talvolta pensiamo che le parole siano interscambiabili o sinonime,

Il *food* lo puoi mettere dentro le scatole che vediamo ormai attaccate a motorini e biciclette per essere consegnato nelle case degli italiani; il cibo puoi anche tentare di metterlo dentro quelle scatole, ma quando ti arriva fa schifo.

dei *rider*, ma una pasta alle vongole o un cibo che caratterizza l'esperienza agroalimentare italiana, se lo infili dentro quelle scatole, perde la sua identità. Purtroppo l'Europa procede e ci vuole portare dentro la *food experience*, dentro l'esperienza del *food*. Noi invece dobbiamo difendere la tradizione del cibo: questa secondo me è la grande sfida culturale che dobbiamo affrontare. Purtroppo, vedo che questo Governo, come quelli passati, nell'innamoramento e nell'ubriacatura europeista, non capisce quello che andiamo a perdere. Non capisce che l'Europa,

ogni tanto sugli insetti, sul vino annacquato e un'altra volta ancora sul latte che arriva da tutt'altro tranne che dal mondo animale. Ebbene, se l'Europa ci porta verso quell'esperienza, non può che essere un'esperienza per noi perdente e fallimentare. Difendere la filiera agricola e agroalimentare vuol dire difendere il nostro patrimonio.

del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della giustizia e il Ministro della salute. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

che fine faranno questo sito e i suoi lavoratori. Ci sono state molte sollecitazioni provenienti dai sindacati e dalle istituzioni locali, ma le risposte non sono adeguate. C'è grande preoccupazione in città e tra le famiglie. Signor Ministro, le chiedo

se non può promuovere un tavolo di confronto con l'azienda, le istituzioni locali e i sindacati, perché stiamo veramente parlando di un pezzo pregiato dell'industria della nostra Nazione,

Il caso non presenta le caratteristiche per essere qualificato come crisi di impresa, bensì necessita, come ribadito dalla stessa Leonardo, di investimenti dedicati per consolidarne la potenzialità di crescita richiesta dal mercato. Ciò anche in ragione del fatto che il settore in cui questa unità opera risulta molto competitivo ed evidenzia la presenza di numerosi operatori di notevoli dimensioni. In tale ottica Leonardo SpA ha riferito che, al fine di garantire automazione la solidità necessaria ad assicurarle una capacità competitiva anche nel medio periodo e dare continuità alle sue attività nel Paese, è stato avviato un percorso per individuare un interlocutore adatto a valorizzarne le competenze e a favorirne lo sviluppo. Tale processo, tuttavia, si trova ancora in una fase preliminare nella quale l'azienda è impegnata a verificare l'eventuale interesse di soggetti terzi che abbiano profilo e attitudine capaci di garantire a questa unità il necessario sviluppo. La stessa si è impegnata a informare tutti gli attori presenti sul territorio degli ulteriori sviluppi, così da assicurare la massima trasparenza e il massimo impegno sull'identificazione delle migliori prospettive industriali dell'unità automazione. È utile rappresentare a tal riguardo che, anche a seguito delle numerose manifestazioni sindacali svoltesi, l'azienda ha comunicato di aver inoltrato apposita comunicazione alle segreterie territoriali e alla RSU (rappresentanza sindacale unitaria), offrendo la disponibilità alla prosecuzione del dialogo relativo all'unità automazione. Naturalmente Leonardo S.p.A. tiene a sottolineare, anche se questo non rileva ai fini del futuro dell'unità automazione, gli importanti investimenti che sull'area di Genova ha precedentemente compiuto e che non sto qui a richiamare. Ritengo che questo percorso, teso a individuare la migliore soluzione possibile, richieda un apposito tavolo. In questo senso, come è stato chiesto anche dalla senatrice Pinotti, questo confronto, che deve preliminarmente svolgersi a livello locale - e in questo senso la prefettura di Genova ha dato la disponibilità a organizzare - dovrebbe coinvolgere tutte le parti sociali e anche le espressioni del territorio. che si tratti di un *player* importante del Paese, legato anche a settori strategici delle nostre industrie in tecnologie avanzate. Pertanto, oltre alla doverosa attenzione nei confronti dei lavoratori coinvolti, c'è anche un aspetto di politica industriale e di strategia che evidentemente il Governo tiene in debita considerazione.

vorrei potermi dilungare un po' di più nella replica, non molto, rimanendo nei tempi. È vero, signor Ministro, non è ancora una crisi di impresa: capisco che rispetto agli strumenti del suo Ministero può rispondermi in questo modo, ma lei ha anche tanta esperienza - quindi posso dirglielo - per sapere che forse non bisogna arrivare ad avere le crisi di impresa. Credo quindi che, nonostante il ruolo che deve avere l'azienda, il Governo possa dare una mano perché non si arrivi a quel punto.

con la ricerca di un *partner* industriale che si impegni a mantenere la qualità del prodotto, a investire su questa qualità in innovazione e ricerca, a mantenere il sito a Genova e i lavoratori.

Ministro, di dare vita a questo tavolo, perché di queste risposte i lavoratori, la città, le istituzioni e, io credo, il Paese

Signor Presidente, signora Ministra, colleghi senatori, com'è noto, la magistratura onoraria sconta da anni una situazione di incertezza che, giunti a questo punto, richiede un'effettiva presa di consapevolezza e di posizione da parte delle istituzioni per ciò che attiene all'individuazione di una soluzione, nel rispetto dei ruoli e del ruolo che i giudici onorari svolgono ormai da anni nel contesto giurisdizionale, che ha persino travalicato tutte le aspettative. Secondo i dati espressi dalle maggiori piattaforme *online* del settore, sono quasi 5.000 i magistrati onorari che operano in Italia e trattano nel complesso circa il 50 per cento solo nel 2019 hanno definito circa 1.100.000 procedimenti. Tutto questo è accaduto evidentemente per una disattenzione del sistema, che ha consentito che la figura del magistrato onorario, che avrebbe dovuto essere l'eccezione, sia diventata invece nel frattempo la regola. Il tema della magistratura onoraria - è stato affrontato anche dalle corti nazionali ed europee, con una serie di pronunzie; da ultimo, addirittura anche dalla Corte costituzionale. Tutte hanno un certo indirizzo, anche se talvolta sono stati enfatizzati gli esiti, oltre quello che era l'effettivo contenuto delle pronunce. Ovviamente però questo ha fatto sì che le stesse associazioni di settore manifestino da tempo una profonda insofferenza, denunciando la necessità che venga attuata una vera e propria riforma del settore, al fine di garantire ai giudici onorari il riconoscimento in termini economici, ma non solo, della loro figura, nonché dello sforzo professionale compiuto, che ha consentito in effetti di tenere in piedi il sistema giudiziario negli ultimi anni. Quindi, di fatto c'è davvero la necessità di una riforma profonda, che metta fine ai contenziosi in atto e soprattutto ne eviti degli altri e, allo stesso tempo, con l'assicurazione della salvaguardia della dignità del lavoro svolto dai magistrati onorari, che oggettivamente va riconosciuto. Quindi, il senso di questa interrogazione è sapere, posto anche l'approssimarsi dall'entrata in vigore della legge Orlando (sarà il 16 agosto 2021), quali siano gli orientamenti del Ministro

Signor Presidente, grazie per il quesito che è stato posto. Il Ministero è al lavoro sul problema della magistratura onoraria. Si è insediata una commissione di studio attualmente è al lavoro sull'analisi delle questioni più rilevanti e sulle criticità emerse nel dibattito pubblico, come ricordate dagli interroganti e sollecitate dalle pronunce delle corti nazionali ed europee. I fronti sono molteplici: c'è un problema di delimitazione delle funzioni; c'è un problema di *status*; c'è un problema di riconoscimento delle tutele del lavoro dei magistrati onorari; c'è un problema delle realtà di chi ha già prestato, nel corso degli anni, questo servizio per lo Stato; c'è da immaginare invece un nuovo futuro per il ruolo della magistratura onoraria. La cornice normativa attualmente in vigore, sulla quale la commissione sta lavorando e sta svolgendo un'attività ricognitiva e di approfondimento, è come noto la cosiddetta legge Orlando, e cioè il decreto legislativo 116 del 2017, che ha inteso realizzare il riordino della magistratura onoraria, declinando uno statuto unico per la categoria. Tale fonte contiene la disciplina relativa al nuovo assetto della magistratura onoraria e, contestualmente, detta disposizioni relative ai magistrati onorari già in servizio al momento della sua entrata in vigore. Ora, la complessità e l'eterogeneità delle posizioni delle varie figure e delle questioni da affrontare ha indotto la commissione da me istituita a suddividersi il lavoro in due sottocommissioni: le problematiche relative ai magistrati onorari in servizio e l'altra studia gli assetti futuri della categoria, valutando altresì le proposte contenute nel disegno di legge all'esame del Parlamento. In questo momento, peraltro, è ancora in corso un programma intenso di audizioni di vari soggetti istituzionali qualificati che possono contribuire a fornire un quadro chiaro sull'analisi delle tutele compatibili con l'incarico onorario svolto. Tra gli altri, i profili allo studio sono la tutela previdenziale, l'indennità omnicomprensiva in relazione all'impegno richiesto ai magistrati onorari, l'impiego nell'ufficio del processo, l'estensione delle competenze da demandare agli stessi. stessi. In questo momento sarebbe prematuro da parte mia esprimere valutazioni sul percorso della commissione, che terminerà i suoi lavori il 25 giugno. Del resto, il prossimo 18 giugno mi risulta che scadrà anche il termine di presentazione degli emendamenti in Parlamento e di cui poi il Ministro terrà conto, insieme ai lavori della commissione. Attendiamo la fine dei lavori. Ribadisco che il Ministero ha come obiettivo principale la funzionalità del sistema giustizia, che oggi appare ancora più urgente in relazione agli impegni assunti con l'Europa. Naturalmente ciò può avvenire soltanto se accompagnato da un'adeguata tutela di tutti gli operatori della galassia giustizia, che sono diversi e numerosi. Qualunque proposta di riforma, peraltro, dovrà seriamente rispettare la cornice dei principi costituzionali ed europei che sono stati enunciati in modo molto preciso da parte della Corte europea, in particolare, e dalla Corte costituzionale, che, da ultimo, nella sentenza n. 41 ha indicato i parametri di riferimento di qualunque intervento normativo in materia, anche ricostruendo il ruolo storico della magistratura onoraria fondamentale, ma distinta rispetto a quella professionale. PRESIDENTE. intervenire in replica il senatore Cucca,

di far ripartire il sistema giustizia nella maniera più adeguata. Il richiamo da lei fatto ai principi costituzionali è veramente importante. Allo stesso tempo, però, ho visto che prende in considerazione gli aspetti principali, e cioè dare dignità a quella funzione di

Credo sia arrivato ormai il tempo di mettere la parola fine alla situazione di incertezza e dalle sue parole mi pare che finalmente i tempi siano considerati maturi. La risposta - ripeto - per me è stata molto soddisfacente e certamente ci sarà necessità di una grande collaborazione fra il Ministero il Parlamento in maniera tale di arrivare alla soluzione migliore e, una volta per tutte, alla fine della situazione di incertezza e precarietà della magistratura onoraria e, allo stesso modo,

L'abuso d'ufficio, che secondo le statistiche dell'ANCI è il reato più gettonato per quanto riguarda la pubblica amministrazione e i sindaci, vede su cento indagini

la complessità normativa, frutto della bulimia eccessiva di questi anni, ha di fatto generato anche lo sforamento in altri settori. ad alcune leggi e anche all'elaborazione giurisprudenziale. Penso al testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro, che rende i sindaci pubblici amministratori responsabili come i dirigenti di qualsiasi società,

ma contiene un mondo. Rispetto a questo mondo, noi le chiediamo, signora Ministro, se non ritenga che, nell'ambito della riforma del processo penale, sia necessario uscire da un feticcio...

l'avviso di garanzia recapitato lo scorso 3 giugno a Stefania Bonaldi, sindaco di Crema, in merito a un incidente che ha riguardato un bimbo che si è schiacciato le dita in una porta tagliafuoco di un asilo comunale; una vicenda che si ricollega - lei lo diceva - a molte altre, che non hanno barriere di appartenenze politiche e sono emerse negli ultimi tempi riguardo la responsabilità penale attribuita ai sindaci quali figure di vertice dell'amministrazione comunale. Siamo di fronte a uno snodo dei più difficili e dei più brucianti che stanno emergendo nel nostro dibattito; uno stato che riguarda il tema di conciliare l'interesse a un costante presidio della legalità e delle responsabilità connesse al rispetto della legge con quello di un'amministrazione scorrevole, che non assuma atteggiamenti difensivi o addirittura fughe, con il rischio di diventare inerte o di paralizzare la macchina pubblica. La legalità va presidiata senza scoraggiare l'assunzione di responsabilità pubbliche. Quando accadono fenomeni come questi, le attività di accertamento delle responsabilità in contesti organizzativi complessi possono richiedere di analizzare i diversi livelli interni all'ente di decisione e di controllo e di svolgere attività investigative che possono coinvolgere una pluralità di soggetti che, a diverso titolo e con poteri, partecipano alla gestione e alla responsabilità, in particolare nel caso da ultimo citato relativo alle questioni inerenti la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, tutti i soggetti devono essere anche tempestivamente assistiti dalle garanzie necessarie per la difesa. Ed è qui, in questo snodo, che talora si verificano situazioni paradossali, perché dal punto di vista giuridico l'iscrizione nel registro degli indagati, l'informazione o l'avviso di garanzia sono istituti processuali posti a tutela della persona attinta dagli atti dell'autorità giudiziaria. Sono istituti di garanzia il loro scopo è assicurare una tempestiva assistenza difensiva, affinché non siano compiuti atti investigativi che riguardano una persona, senza che questa ne sia a conoscenza e possa essere assistita dal difensore. però che, nei fatti, la comunicazione all'interessato dell'avviso di garanzia spesso diventa di pubblico dominio e rischia di innescare un meccanismo di stigma sociale, a detrimento anziché a vantaggio della persona destinataria. Questo è un nodo a cui sono molto sensibile ed è quello di restituire ai fondamentali passaggi dell'iscrizione della notizia del reato e della comunicazione che ne viene fatta all'indagato il significato di tutela che gli è proprio. due osservazioni, una sul diritto vigente e una sui lavori che sta svolgendo la commissione in materia di processo penale. Invero, nel diritto vigente, già oggi l'articolo 335 prevede che l'iscrizione nel registro deve essere riferita alle persone alle quali il reato è attribuito e che quindi dovrebbero già essere individuate come possibili responsabili della commissione del reato. La commissione Lattanzi, che ha lavorato sulle riforme del processo penale, ha previsto una direttiva, all'articolo 3, che dovrebbe riguardare i presupposti dell'iscrizione, peraltro già in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale richiede specifici elementi indizianti e non meri sospetti per l'iscrizione nel registro. Nella relazione si legge che i criteri di delega sono volti a «precisare i presupposti per l'iscrizione nell'apposito registro della notizia di reato e del nome della persona a cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza, uniformità delle iscrizioni» e «prevedere che la mera iscrizione del nominativo della persona non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo». Credo che anche la questione del tempo, del momento in cui debba avvenire questa iscrizione, sia delicata: debbono esserci specifici elementi indizianti... Mi fermo qui, ma sappiate che questo tema è all'attenzione e sarà affrontato anche nel pacchetto delle riforme, che speriamo possa arrivare al più presto all'esame del Parlamento e che abbiamo elaborato negli ultimi mesi.

45 e, nell'incertezza, sceglie il modello 21: iscrizione della notizia di reato a carico di persone note. Da qui inizia il circuito mediatico-giudiziario. Credo che il problema oggi non sia quello della separazione delle carriere, ma sia estendere

*(FdI)*. Signor Ministro, oggi vorremmo occuparci della enorme massa di prestazioni che compongono un compendio di sanità sospesa o sanità negata, in alcuni casi drammaticamente I numeri sono noti: da gennaio a settembre 2020 sarebbero state perse 52 milioni di visite specialistiche e diagnostiche;

per non parlare dell'allarme sulle patologie psichiatriche. Rispetto a questi numeri potevamo fare meglio? Potevamo organizzare meglio tutta la vicenda dell'emergenza? Questo lo vedremo *a posteriori.* Oggi

Ministro, di quel mezzo miliardo che abbiamo stanziato nel decreto-legge agosto e che le Regioni hanno ricevuto con l'impegno di utilizzarlo entro il 31 dicembre? Senza avere contezza di come è stato usato quel denaro,

inutile mettere danaro per le assunzioni, se i concorsi restano deserti, perché non ci sono professionisti. Pertanto, al di là del mettere danaro, che comunque è un'operazione assolutamente utile e opportuna, bisogna capire quali sono gli intendimenti per agire in modo reale su questo enorme problema.

Signor Presidente, ringrazio i senatori interroganti che mi offrono l'opportunità di toccare un tema di particolare importanza; d'altronde su questa materia abbiamo già avuto modo di di confrontarci anche proprio con il senatore Zaffini. Non vi è dubbio che la lettura comparativa dei dati relativi agli anni 2019 e 2020, pur tenendo conto di una costante contrazione dei ricoveri ospedalieri che in verità è in atto già da diversi anni, con un tasso di ospedalizzazione che è sempre stato in calo dal 2001 ad oggi, evidenzia una fortissima flessione dell'erogazione complessiva dei ricoveri nel 2020. Porto solo il dato relativo ai ricoveri: una perdita in termini di volumi di 1.301.048 prestazioni, attribuibile senza dubbio all'impatto della pandemia sugli assetti organizzativi della nostra offerta sanitaria. In considerazione degli effetti sulla salute di una così ampia riduzione dell'erogazione delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, è indispensabile mettere in atto efficaci strategie per il completo recupero, riprogrammando adeguatamente e tempestivamente l'attività ospedaliera e ambulatoriale, alla luce del miglioramento delle condizioni organizzative legate all'aumento della copertura vaccinale nel personale sanitario e nella popolazione generale. Il Ministero della salute - come lei ricordava - con il decreto-legge agosto ha affrontato questa questione, promuovendo un finanziamento straordinario di circa mezzo miliardo, mettendolo a disposizione delle Regioni. Quanto, in particolare, all'impegno delle risorse previste nel decreto-legge, il Ministero della salute ha ricevuto da tutte le Regioni il piano operativo regionale di recupero di quelle liste d'attesa. Ciascun piano, conformemente a quanto stabilito dalla legge, prevede un modello organizzativo strutturato sulla base delle esigenze territoriali, nonché delle prestazioni perse a causa dell'emergenza pandemica.

Quindi, è chiaro che le risorse che dovevano servire per recuperare il pregresso, in realtà, per larghissima parte, non sono state utilizzate, perché le strutture sanitarie non hanno potuto recuperare il passato, ma hanno dovuto nuovamente - come già avvenuto in primavera - rioccuparsi dell'emergenza pandemica. Sulla base di questa valutazione nel decreto-legge sostegni-*bis* abbiamo inteso estendere la durata dell'intervento straordinario già fatto per tutto l'anno successivo, cioè il 2021. Chiaramente è anche previsto il coinvolgimento degli erogatori privati - questa è una differenza tra le due norme - al fine di rendere più efficace il piano di interventi. Il Ministero, inoltre, parallelamente all'azione di monitoraggio già intrapresa, ha chiesto a ciascuna Regione una puntuale relazione sullo stato dell'arte e sulle criticità riscontrate, che saranno oggetto interventi. In conclusione, questo sarà il tema più importante per il nostro Servizio sanitario nazionale nei prossimi mesi, perché il mezzo miliardo, per quanto mi riguarda, è solo il primissimo pezzo di un impegno a cui dovremo sicuramente attenerci in maniera molto forte.

a interloquire nei prossimi mesi per tutte le patologie oncologiche e cardiologiche. L'aver sospeso i *follow-up* oncologici determinerà evidentemente un problema gigantesco, che non possiamo affrontare semplicemente rimettendo un po' di denaro. Ripeto: il danaro è condizione indispensabile, ma certamente non sufficiente. Servono provvedimenti di sistema. Faccio un banale esempio: sappiamo perfettamente che oggi è necessaria una riforma profonda delle scuole di specializzazione e serve poter utilizzare gli specializzandi

Non agire sul personale renderebbe inutili anche tutte le misure contenute nel PNRR e nel progetto di riforma della sanità territoriale,

più alcun alibi. Se il Covid è stato un alibi, una scusa, un motivo, oggi non ne abbiamo più. Oggi abbiamo un'enorme massa di prestazioni sanitarie arretrate, che si aggiunge a un problema cronico di disuguaglianza di somministrazione dei LEA tra Nord e Sud, che dobbiamo non affrontare, Su tutto questo, Ministro, ci aspettiamo qualcosa di assolutamente diverso, ma soprattutto di rapido e immediato.

salute* - Premesso che: le vaccinazioni anti COVID stanno procedendo a ritmi sostenuti e l'adesione massiccia dei giovani suscita grande soddisfazione; se è vero che i vaccini sono tutti efficaci, non sono tutti uguali; il vaccino Astrazeneca può causare una trombosi venosa associata a diminuzione delle piastrine, che si presenta a distanza di 5-15 giorni dalla vaccinazione e può avere esito fatale. Questa complicanza è stata descritta in soggetti dai 20 ai 55 anni, ma le persone di gran lunga più colpite sono le giovani donne. La trombosi piastrinopenica da vaccino, che non è provocata dai vaccini a RNA, è molto rara. Ovviamente però in una vaccinazione di massa anche una complicanza molto rara, ma potenzialmente letale, può causare un numero significativo di morti, anche in soggetti che, per sesso ed età, come le giovani donne, hanno un rischio praticamente nullo di morire di COVID; sono molte le voci autorevoli (Gruppo medici volontari vaccinatori di Genova, le Scienziate per la Società, l'associazione Luca Coscioni, Le Scienziate per la Scienza, GIMBE e singoli autorevoli medici e scienziati) che hanno lanciato un appello

Chiedo quindi al Ministro di sapere quali azioni intenda porre in essere affinché vengano bloccati o almeno riparametrati gli *open day* AstraZeneca, attualmente senza restrizioni di età, per non mettere in ulteriore pericolo le fasce giovani che tanto hanno sofferto in questa pandemia e non devono ulteriormente pagare, soprattutto le giovani donne; quali azioni intenda intraprendere affinché la volontà di riprendere una vita sociale come era prima della pandemia, che i giovani aspirano tanto a riprendere, non sia maggiore della consapevolezza dei rischi che si corrono nell'effettuare il vaccino AstraZeneca.

concludendo comunque che i benefici del vaccino restassero complessivamente superiori ai rischi e che gli eventi trombotici venosi in sedi inusuali associati a livelli bassi di piastrine dovessero essere elencati come effetti indesiderati molto rari. L'EMA ha inoltre raccomandato che l'uso di AstraZeneca durante le campagne di vaccinazione a livello nazionale tenesse conto della situazione pandemica e della disponibilità dei vaccini nelle singole Nazioni.

sulla base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte dell'elevata mortalità da Covid-19 nelle fasce di età più avanzate. Successivamente, a fine aprile, su richiesta della Commissione europea, l'EMA ha concluso un'ulteriore valutazione analizzando i benefici e i rischi del vaccino nelle diverse fasce di età e in diversi scenari epidemiologici, alla luce dei tassi di infezione mensili. L'esito ha dimostrato che i benefici della vaccinazione aumentano con l'aumento dell'età e del livello di circolazione del virus. Tali dati sono stati ulteriormente valutati dall'Aifa ed è stato ribadito che il profilo beneficio-rischio risulta progressivamente più favorevole all'aumentare dell'età. L'effetto è tanto più marcato in una condizione di diminuita incidenza dell'infezione in quanto vengono a ridursi i rischi di malattia grave Covid-19. Voglio ricordare che l'Italia è passata nelle ultime settimane da un livello di circolazione alto ad uno medio ed ora è ad uno basso. Queste valutazioni saranno sicuramente considerate nel prossimo parere del CTS. Mi permetta però di ricordare sempre che i vaccini sono la vera arma di cui disponiamo per chiudere questa stagione così difficile e che tutti quelli approvati da EMA e Aifa sono sicuri ed efficaci. La campagna di vaccinazione nel nostro Paese ha superato le 40 milioni di dosi somministrate: è un risultato molto incoraggiante che sta producendo un esito positivo in termini sia di riduzione dei contagi che della mortalità e della pressione sui nostri servizi sanitari. nuova finestra") *(Misto)*. Signor Ministro, le ricordo che il primo scopo di un atto medico è sempre il beneficio, almeno probabilistico, del paziente. Il beneficio della popolazione è un vantaggio aggiuntivo che non può essere conseguito a danno del paziente, Non dimentichiamo che il vaccino ha ancora un'autorizzazione di emergenza. I dati aggregati ci suggeriscono che la valutazione rischio-beneficio debba essere fatta per sesso e per fascia di età. La medicina di genere è sempre stata trascurata nel nostro Paese e poco si dà attenzione alle donne in risposta a un trattamento medico. Questo è un caso che io considero particolarmente grave: aver trascurato cioè i dati aggregati sulle giovani donne. Anch'io - la mia storia lo dice - penso che i vaccini siano un'arma formidabile, ma tutta questa storia ha minato profondamente la fiducia dei cittadini e quindi chiedo al Ministro una maggiore autorevolezza nel limitare l'uso di AstraZeneca nelle giovani donne, al fine di poter riacquistare la fiducia e di proteggere la popolazione più giovane del nostro Paese, affinché in futuro tutti aderiscano con grande fiducia alle vaccinazioni. Questo forse è stato un caso sfortunato in cui non si è conquistata la fiducia dei cittadini, ma sono convinta che lei possa apportare una rapida

*(L-SP-PSd'Az)*. Signor Ministro, lei saprà bene che l'8 aprile di quest'anno l'Assemblea del Senato ha approvato a stragrande maggioranza, con la firma di tutti i Gruppi, una mozione con la quale si chiedeva di aggiornare i protocolli e le linee guida sulla presa in carico dei pazienti pazienti che soffrono di Covid-19, tenuto conto delle esperienze che i medici hanno messo in campo.

direttamente i pazienti. La domanda è perché si sia optato per questa testarda quanto ingiustificata insistenza su un protocollo di vigile attesa e tachipirina, a sfavore, in molti casi, di efficaci cure precoci e domiciliari. La domanda è molto semplice: perché?

e ritengo che la circolare gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars Covid del 26 aprile fornisca indicazioni univoche in merito alla gestione in ambito domiciliare dei pazienti affetti da forme lievi di Covid-19 su diversi aspetti, quali l'identificazione dello stato clinico della malattia, l'identificazione della classe di rischio del paziente, gli strumenti di monitoraggio delle condizioni critiche, le modalità di monitoraggio della saturazione dell'ossigeno, i sintomi di allarme, i principi di gestione farmacologica. Tali indicazioni, proprio perché da applicarsi al domicilio del paziente, valgono uniformemente sul territorio nazionale, prescindendo dal modello organizzativo regionale. Le raccomandazioni della terapia farmacologica fornite all'interno della circolare riflettono, a differenza di quanto affermato, le indicazioni emanate dall'Aifa, formulate tenendo conto di studi nazionali ed internazionali e confermate dalle evidenze emerse dalle revisioni sistematiche della letteratura e conformi a quanto suggerito dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, da ultimo nelle raccomandazioni pubblicate e divulgate dall'OMS nel documento «*Therapeutics*and **COVID*-*19*: *living guideline».** Sulla necessità di un lavoro in *team* multidisciplinare e multiprofessionale attraverso il confronto e la condivisione di specifiche competenze, ribadisco che la circolare in oggetto è stata redatta da un gruppo di lavoro multidisciplinare costituito da tutti i rappresentanti delle istituzioni, proprio a partire dalle sigle che lei ha indicato, del mondo scientifico e delle professioni, dotati tutti di elevata competenza ed esperienza, che ha lavorato all'aggiornamento della precedente circolare del 30 novembre 2020, con l'obiettivo di fornire indicazioni operative alla luce delle nuove conoscenze acquisite e delle esperienze intervenute sia in ambito farmacologico che clinico, tenendo conto delle indicazioni dell'Aifa sui singoli trattamenti farmacologici e dei pareri del Consiglio superiore di sanità. Nella medesima circolare è stato inoltre inserito un riferimento importante alle prestazioni in telemedicina. Sulla necessità di rafforzare l'assistenza domiciliare, credo che questo Governo sia sempre molto impegnato, in piena sintonia con l'Istituto superiore di sanità, il Consiglio superiore di sanità, Aifa e Agenas.

l'intervento che stiamo predisponendo nel PNRR arriveremo a essere il primo Paese d'Europa per assistenza domiciliare, con il 10 per cento. Oggi i migliori modelli in Europa sono Svezia e Germania,

*(M5S)*. Signor Ministro, grazie allo straordinario patrimonio di competenze operanti presso 50 registri tumori di popolazione e 7 registri specializzati del capillare assetto organizzativo nel territorio, i registri tumori italiani hanno garantito elevati *standard* di qualità al dato epidemiologico sulla patologia oncologica. Il 22 marzo 2019 veniva approvata la legge n. 29 sull'istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Tale legge, oltre alla raccolta, all'analisi e alla pubblicazione di dati epidemiologici generali, mira alla sorveglianza epidemiologica, oncologica e infettivologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo. È chiaro il riferimento all'importante ruolo che potrebbe essere rivestito dalla predetta norma anche nell'attuale pandemia Covid, in riferimento ai soggetti fragili portatori di malattia oncologica. Nello specifico, l'articolo 1, comma 2, prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento da adottare su proposta del Ministero della salute, siano individuati i dati e le modalità relative al loro trattamento, nonché i soggetti da inserire all'interno della suddetta Rete, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati, garantendo in ogni momento agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dai regolamenti europei in materia di *privacy,* razionalizzando gli obblighi informativi, in armonia con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, nell'ambito di un sistema integrato e unico di flussi di dati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie. Il Ministero della salute può inoltre stipulare accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che, da almeno dieci anni, operino senza fini di lucro nell'ambito dell'accreditamento del sistema di rilevazione. Alla data odierna, i decreti non hanno trovato piena attuazione e chiediamo quindi di sapere:

ad individuare le relative risorse, il personale, nonché le infrastrutture materiali e immateriali per supportare le attività del registro; se e quali formali interlocuzioni siano state avviate con soggetti aventi i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 6, della legge quali iniziative si intenda assumere per non disperdere e per preservare lo straordinario patrimonio di competenze operanti presso i registri tumori italiani; se e come si intendano conferire nell'istituendo

chiarire una vicenda particolarmente importante. Per rendere operativo il registro nazionale tumori previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, il Ministero della salute, coinvolgendo anche esperti esterni all'amministrazione e responsabili dei registri regionali e referenti dell'Associazione italiana dei registri tumori ha attivato un apposito gruppo di lavoro interdisciplinare che ha predisposto un testo di regolamento. La successiva adozione della legge n. 29 del 2019 ha richiesto una riflessione approfondita per scongiurare il rischio di duplicazioni di banche dati sanitarie.

Per evitare di rallentare il raggiungimento degli importanti obiettivi informativi, statistici e sanitari in gioco, si è ritenuto di proseguire con la predisposizione dello schema di regolamento del registro tumori nazionale e del relativo disciplinare tecnico, che potrà successivamente e auspicabilmente confluire, insieme agli altri registri e sistemi di sorveglianza, nel più ampio contenitore della Rete nazionale, la cui regolamentazione non potrà che seguire logicamente e cronologicamente quella dei singoli registri e sistemi di sorveglianza. Lo schema di regolamento del registro nazionale tumori è già stato sottoposto per una valutazione preliminare al Garante per la protezione dei dati personali, che ha fornito utili suggerimenti, validi anche per la regolamentazione degli altri registri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2017. È stata inoltre già predisposta la richiesta del prescritto parere preventivo del Consiglio superiore di sanità. Ciò premesso, con riferimento alla richiesta di conoscere la sede fisica del registro nazionale, rappresento che, in coerenza con il menzionato decreto il registro sarà ospitato dall'infrastruttura tecnologica del Ministero della salute. In particolare, la realizzazione, la gestione operativa e lo sviluppo saranno affidati alla direzione generale competente in materia di sistema informativo e statistico sanitario, che acquisirà per i profili sanitari il parere della direzione generale competente in materia di prevenzione. Mi preme inoltre evidenziare che è intenzione del Ministero non disperdere lo straordinario patrimonio di dati finora raccolti nei registri tumori italiani, valorizzare le competenze di esperti esterni e di Airtum e preservare il capillare assetto organizzativo, come dimostrato dal fatto che, nell'emanando schema di regolamento, si dispone che le Regioni realizzino il proprio registro tumori, tenendo conto dei registri al momento operativi. Infine, con riguardo alle risorse, voglio fornire rassicurazioni sul fatto che un finanziamento per l'implementazione del registro nazionale è previsto nell'ambito dell'attuazione del PNRR e che per i registri regionali è in corso di adozione il decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di riparto degli appositi fondi destinati dalla legge n. 160 del 2019.

qualsiasi decreto che voglia comunque centralizzare le attività della registrazione dei casi di patologie oncologiche deve necessariamente preservare l'autonomia dei singoli registri, registri, passando dal filtro del coordinamento regionale e rendendo i dati del registro tumori nazionale non sottoposti a sistemi autorizzativi, con lo scopo di evitare una deriva burocratica e di favorire la sorveglianza epidemiologica della patologia oncologica. Per questo auspichiamo che vengano individuate al più presto le risorse e le infrastrutture per supportare le attività del registro tumori nazionale e della Rete nazionale dei registri tumori. che le modalità di utilizzo del dato epidemiologico siano disciplinate da un comitato tecnico-scientifico, con competenze specifiche nella registrazione della patologia oncologica, nella sorveglianza epidemiologica e nella prevenzione dei tumori. Accogliamo con piacere la comunicazione in merito alla collaborazione già in atto con Airtum e con tutte le società scientifiche che hanno già mostrato grande esperienza sul tema e la ringraziamo.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

gentili colleghi e gentili colleghe, sono passati cinque anni dall'ultima decisione del Comitato economico e sociale europeo, che denunciava come l'Italia stesse violando la Carta sociale europea. Ma il verdetto è sempre quello: in Italia permangono disparità di accesso all'interruzione di gravidanza a livello locale e regionale e i dati forniti dal Governo non dimostrano che il personale medico specializzato nel fornire il servizio sia sufficiente. Il Comitato ha notato che, sulla base degli ultimi dati disponibili, risalenti al 2018, il numero di ginecologi obiettori di coscienza, invece di diminuire, è aumentato e che vi è una disparità di accesso a livello regionale, che porta almeno il 5 per cento delle interruzioni di gravidanza a essere eseguite in Regioni diverse da quella dove vive la donna. Dopo oltre quarant'anni dalla promulgazione della legge n. 194, che riconosce alle donne il diritto di interrompere la gravidanza entro il primo trimestre, c'è ancora chi propone la sua sospensione o, peggio, la sua eliminazione, minando i diritti sessuali e riproduttivi di noi donne. È così che ci ritroviamo ancora oggi a prendere coscienza di come per molte donne italiane questo diritto sia un rischio, a raccontare quanto sia difficile l'aborto in Italia. Come denuncia anche la Laiga (Libera associazione italiana ginecologi per l'applicazione della legge 194), secondo la relazione ministeriale del 2018 solo il 59,6 degli ospedali pratica l'interruzione di gravidanza; la maggior parte di questi la fa entro i novanta giorni. L'interruzione nel periodo successivo, per grave rischio alla madre alla madre o malformazione grave del feto, non viene fatta nella maggior parte degli ospedali italiani. Sono ancora molte, troppe le donne che, oltre ad affrontare una decisione estremamente difficile come quella di un'interruzione di gravidanza, devono scontrarsi con questa dura realtà, che di fatto, come i come i dati descrivono, non permette alle donne di esercitare un diritto di legge che è stato loro riconosciuto. Tra le Regioni in cui l'aborto non è c'è anche l'Umbria, che ha prima eliminato la possibilità di farlo in *day hospital*, per poi fare un passo indietro dopo le nuove linee guida al riguardo del Ministero della salute. Proprio così: la Giunta regionale dell'Umbria, in piena emergenza Covid, ha provato a cambiare le carte in tavola. Ma non solo in Umbria; anche in altre Regioni non c'è la possibilità di effettuare l'aborto...

Signor Presidente, da siciliana tengo a chiarire un aspetto che riguarda la mia Regione. Spesso si dice che la Sicilia è fallita. No, la Sicilia non è fallita; è il governo regionale a essere fallimentare. La crisi più visibile dai cittadini riguarda proprio i Comuni e si tratta di una crisi stratificata e datata, conseguenza quasi esclusivamente del comportamento delle altre istituzioni pubbliche coinvolte a vario titolo. È nella gestione degli enti locali siciliani. L'attuale governo regionale, all'atto del suo insediamento, avrebbe dovuto accertare le risorse finanziarie sottratte dallo Stato alla Regione Siciliana. Si è trattato di immotivata erosione, come denunciato periodicamente della Corte dei conti siciliana, non consentendo ai Comuni di soddisfare i fabbisogni primari della popolazione. L'inerzia del governo regionale, unitamente ai dispiegati silenzi di altre istituzioni pubbliche, ha condotto all'attuale crisi finanziaria del comparto delle autonomie locali siciliane. A ciò aggiungasi l'impegno del governo regionale a non rendere efficiente e funzionale la riscossione fiscale in Sicilia, una riscossione che dovrebbe essere anche al servizio dei Comuni siciliani.

Non sarà la postergazione dei termini di approvazione dei documenti contabili e, quindi, il governo della Regione Siciliana deve essere in grado di definire, anche delegando l'attività a soggetti e strutture competenti, competenti, con lo Stato un accordo che liberi immediatamente le risorse finanziarie necessarie per i Comuni siciliani. Si tratta dell'avvio di un'attività che dovrà concludersi con la completa estinzione del debito dello Stato nei confronti della Regione Siciliana. Se sono in crisi i Comuni siciliani è utopistico pensare all'applicazione del *recovery plan* in Sicilia, considerato infine che si tratta di interventi *post* pandemici e, dunque, aggiuntivi e non sostitutivi. Occorre, dunque, verificare preliminarmente l'applicazione dell'articolo 38 dello Statuto e della legge n. 17 del 2018.

concessione autostradale sulla Brescia-Padova di cui è proprietario Atlantia, dei fratelli Benetton, così meritori nell'aver gestito le autostrade italiane, tanto da far crollare il ponte Morandi per carenza di manutenzione, che si è trasformato in utili per gli azionisti, in lutto per le famiglie e disastro per il Paese e, in particolare, per la città di Genova. Segnalavo che questa estensione era fatta da questo dirigente del Ministero delle infrastrutture sulla base - esplicitamente citata - di una deliberazione del Comitato che ha un piccolo problema: un anno prima della firma di quel dirigente del Ministero e, cioè, il 21 gennaio del 2019 quella deliberazione era stata definitivamente annullata dal Consiglio di Stato. Gli interessati hanno anche fatto ricorso alla Corte di cassazione che li ha respinti ritenendo addirittura inammissibile la loro richiesta. Mi aspettavo da parte del Ministro un ringraziamento per aver segnalato una cosa che fa regalare dallo Stato su una struttura di sua proprietà alla solita Atlantia della famiglia Benetton la bellezza di un 1.158.000 al giorno. Pertanto, da quando io ho fatto la segnalazione, già sono stati regalati altri 113 milioni alla famiglia Benetton, il risparmio di due anni per il famoso taglio dei parlamentari. parlamentari. Nei tre minuti in cui sto parlando saranno 2.414 gli euro regalati a questa azienda e saranno 2,5 miliardi fino al 2026. Bene: io non ho ricevuto ringraziamenti dal Ministro - pazienza - ma neanche l'ombra di una risposta. L'interrogazione

recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19»